Comunico che in data 28 ottobre è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della giustizia:* «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»

al Parlamento francese, alla città di Nizza e, ovviamente, alle vittime di questo nuovo, gravissimo attentato terroristico. Pochi minuti fa, alcuni terroristi hanno colpito la città di Nizza, assassinando e decapitando tre cittadini che erano in preghiera nella cattedrale di Notre-Dame. Non si ha ancora contezza di quante siano effettivamente le vittime, si ha la certezza, per quanto ha dichiarato anche il sindaco che si tratti di un attentato terrorista e che almeno uno degli aggressori sia stato colpito ed arrestato. del secondo recente episodio che colpisce la Francia: quindici giorni fa è stato assassinato e decapitato un professore che aveva osato insegnare la libertà di espressione nella scuola francese. La scuola e la chiesa, gli emblemi della nostra civiltà, sono state colpite nel cuore della Francia: quindici giorni fa, nella periferia di Parigi, e questa mattina, nel centro di Nizza. Ricordo a noi tutti che quest'ultima è già una città martoriata,

esprimere all'Assemblea nazionale francese e al popolo francese la nostra solidarietà, nella consapevolezza che l'attacco ripetuto alla Francia e ai simboli della nostra civiltà - la scuola e la libertà di espressione, la chiesa e la libertà di religione - sia un attacco a tutti noi, italiani ed europei, che pertanto che pertanto dobbiamo tutelarli fino in fondo. Non sfugge ad alcuno che questo sia accaduto pochi giorni dopo che una persona, che ho difficoltà a nominare come presidente e anche come signore, cioè Erdoğan, aveva soffiato sul fuoco, aizzando il fondamentalismo islamico, di fatto, a difendersi, quindi a colpire nel cuore d'Europa. Questo è inaccettabile e noi, come Parlamento e come Governo, le necessarie conseguenze.

a pochi minuti dall'attacco nella cattedrale di Nizza per esprimere sconcerto e sgomento, in un momento così drammatico per la storia del pianeta,

di questo nuovo attentato terroristico. Vogliamo essere vicini al popolo francese e alle sue istituzioni. La dinamica, almeno secondo le prime notizie, fa pensare a un attentato di matrice islamista,

a due settimane - come ricordava il collega Urso - da quella dell'insegnante Samuel Paty, decapitato a Parigi per aver parlato agli studenti delle vignette di «Charlie Hebdo». Anche a Nizza una donna sarebbe stata decapitata e uno degli assalitori è stato ferito e fermato polizia. Stiamo vivendo un momento drammatico per la pandemia, questo nemico invisibile che sta mietendo migliaia e migliaia di vittime e causando sofferenze nel mondo.

classiche. Ecco perché in troppi su questo pianeta stanno soffiando sul fuoco. Occorre abbassare i toni:

innanzitutto, a nome del Gruppo Lega, porgo le mie condoglianze e il mio cordoglio al popolo di Francia, alle istituzioni francesi e, in particolare, alla comunità cristiana francese. Nel dicembre di due anni fa, in quest'Aula, da questo posto, intervenni

e sempre con lo stesso scopo, ovvero colpire le radici identitarie del popolo francese, nella loro declinazione cristiana. Se ci riteniamo laicizzati

che ritengono la dimensione spirituale assolutamente attuale e immanente alla realtà politica. Anzi, affermare valori religiosi (che non condividiamo,

che esiste solo per noi, ma non per loro; sono lodati dalla loro popolazione e sono considerati eroi e, tra l'altro, non ci sono *imam* che li condannino, perché non possono farlo, in quanto eseguono quanto previsto dal Corano e dagli *hadith* del profeta Maometto. quindi un appello al Governo a considerare la sicurezza del nostro Paese. Bene lavorano i nostri servizi di *intelligence*: mi raccomando, continuiamo a supportare l'azione dei nostri servizi di sicurezza, tenendo presente l'obiettivo del nostro nemico, che non è quello di una classica politica di potenza.

alla città di Nizza, all'Assemblea nazionale e al popolo francese. La dinamica dell'assalto e le testimonianze lasciano pochi dubbi sulla matrice e sull'estrazione politico-culturale di questi assassini, che tuttavia, al di là del singolo episodio, ci episodio, ci richiamano, come cittadini europei e italiani, a una presa di coscienza sull'eccezionalità della situazione che stiamo vivendo,

è naturale purtroppo che malintenzionati o anche gruppi politici organizzati prendano iniziative per lacerare lo spirito unitario che un popolo deve avere in questo momento e per seminare paura e terrore. Da qui l'appello che, ancora una volta, rivolgo a nome del MoVimento 5 Stelle a tutte le forze politiche. Davanti alle difficoltà dei cittadini e all'esasperazione, l'appello è al massimo dell'unità politica, al di là delle differenze, e a una leale collaborazione repubblicana, che è la sola che in questo momento ci consente di fare tutti gli sforzi necessari per fronteggiare e rispondere alle esigenze dei cittadini. Al contempo, occorre lanciare un messaggio a chi volesse seminare terrore e paura e destabilizzare: la democrazia in Italia è un bene prezioso che tutti, a partire dalle forze politiche presenti in quest'Aula, lealmente e insieme, siamo pronti a difendere con tutti i mezzi necessari. *(Applausi)*.

al presidente Macron, all'Assemblea nazionale francese e a tutti i cittadini francesi, colpiti in questo momento da un tragico avvenimento. È chiaro che gli accertamenti sono in corso e bisognerà verificare

valori del rispetto e della tolleranza reciproca. Signor Presidente, mi unisco agli interventi dei colleghi su quanto è successo solamente pochi minuti fa nella città di Nizza, in uno dei luoghi simbolo di quella città, della Francia, della nostra Europa, la cattedrale di Notre-Dame. Un orrore indicibile, Presidente, che però noi abbiamo il dovere di affermare e di denunciare in questa Aula. L'omicidio, la decapitazione

facciamo i conti e siamo alle prese con gli effetti della terribile pandemia che compromettono e mettono a dura prova la tenuta sociale ed economica dei nostri Paesi. In tale contesto, l'attentato di questa mattina ha l'obiettivo di creare paura, disorientamento irrazionalità. A tutto questo la politica deve rispondere con la massima fermezza. Esprimo solidarietà, a nome del Partito Democratico, alla Repubblica francese, al popolo francese e alla città di Nizza, già colpita da un terribile attentato terroristico nella sera del 14 luglio 2016, durante i festeggiamenti di popolo per celebrare di questa mattina è un tentativo innanzitutto di minare lo Stato di diritto. A questo si risponde rafforzando lo Stato di diritto e dimostrando

è il culmine di una sequenza che ha colpito in questi anni l'Europa, in particolare la Francia, e che ha visto solamente pochissimi giorni fa,

vicenda di gravità inaudita. Quell'omicidio voleva colpire anch'esso il simbolo dello Stato di diritto, l'insegnamento e l'educazione alla laicità e alla libertà. che la fermezza che noi dobbiamo assumere di fronte a tutto questo si debba esprimere non solo nello sdegno di questa Aula stamattina, ma in una risposta molto forte. Chiedo allora, per suo tramite, che quest'Aula possa dedicare alla figura di Samuel Paty, così simbolica, un'apposita sessione di lavoro per riaffermare l'importanza dei valori di libertà e di laicità

Presidente, il Gruppo per le Autonomie esprime solidarietà alla famiglia e al popolo francese per il drammatico e orribile attentato Vorrei qui brevissimamente ricordare la frase di Muhammad Ali, che è il nome che Cassius Clay prese dopo essersi convertito all'Islam: all'Islam: «L'Islam non è odio. Dio non sta con gli assassini». È una sintesi perfetta e sublime. No al fanatismo, no a chi lo coltiva, no chi lo usa come uno strumento di lotta politica. La responsabilità della politica è riuscire ad essere altro rispetto all'odio e alla violenza che ne scaturisce. Dobbiamo essere capaci di dimostrarlo e all'altezza di questa sfida, anche qui, noi, oggi. Questa e solo questa è la responsabilità della politica.

al popolo francese, alle sue istituzioni, alla città di Nizza in particolare, già colpita anni fa, e alla Francia, colpita diverse volte da questo tipo di terrorismo. Sulla natura di questo terrorismo credo che non ci possano essere dubbi, considerate le modalità con cui ha agito l'assassino, che, da quanto si sa, era isolato (ma non lo sappiamo ancora con certezza). ciò che ha gridato durante e dopo aver commesso i suoi omicidi, com'è stato più volte testimoniato, invocando il suo dio, è evidente la matrice: non è terrorismo generico, ma islamico. Di fronte a questo dobbiamo avere un atteggiamento, sì, laico, com'è stato detto, ma ciò significa essere fedeli ai valori della nostra Costituzione,

solidarietà, ricordandosi però che non ci si può limitare ad essa e a un'esecrazione generica. Bisogna andare nel concreto e colpire chi incita all'odio e diffonde questo tipo di ideologia. La condanna e il cordoglio unanime espressi ora in Aula da tutti i Gruppi mi consentono, a nome della Presidenza e di tutto il Senato, di invitare

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 1721 e dei

Signor Presidente, oggi siamo chiamati a votare la legge di delegazione europea 2019-2020, presentata in Senato già nel febbraio scorso e accompagnata da un attento esame dei suoi quasi 30 articoli; un esame su materie particolarmente significative, che ci era sembrato superato dal lavoro a cui ci ha costretti l'emergenza sanitaria, che ha stravolto e continua a stravolgere la vita sociale, economica e politica in tutto il mondo. un lavoro contestuale non facile, quello sul tavolo nazionale ed europeo, per l'adozione di strumenti efficaci a contrastare gli effetti prodotti dalla pandemia in termini di tutela della salute, ma anche di contrazione economica e di aumento del debito pubblico, delle disuguaglianze e delle disparità territoriali. Purtuttavia, proprio la legge di delegazione europea rappresenta uno strumento fondamentale per il processo di armonizzazione e avvicinamento degli ordinamenti dei singoli Stati membri, che quindi contribuisce a realizzare un'Unione sempre più stretta per un progetto che riteniamo non solo possibile, ma dovuto, l'orizzonte di un destino comune. La crisi sanitaria ha dimostrato quanto sia importante essere parte di un'Unione capace di mettere in campo propri strumenti di sostegno, dallo state supported short-time work (Sure), all'intervento della BEI e della BCE. In questo contesto, la legge di delegazione europea 2019-2020, che consente l'adeguamento a ben 33 direttive europee e 14 regolamenti, qualificherà la nostra partecipazione a quel processo d'integrazione europea. Anche su questo ci giochiamo la nostra credibilità, credibilità, da mettere certamente in campo nel far fronte all'emergenza sanitaria, ma anche nella definizione della strategia di ripresa e resilienza e per l'impiego dei 208 miliardi del Next generation EU, risorse faticosamente negoziate, ma che rischiano - ahimè - di essere messe in discussione da quei Paesi sovranisti che fanno fatica a condividere non solo le spinte europeiste, ma anche il patrimonio culturale e democratico di difesa dei diritti fondamentali e delle libertà comuni, un lavoro parallelo tra l'attuazione delle norme europee e la realizzazione delle riforme strutturali indicate nell'ambito del semestre europeo, che dovrebbero contribuire a superare la crisi, ma anche le tante storture che hanno frenato da anni crescita stabile e qualità dello sviluppo, dunque riforma della giustizia e del sistema della pubblica amministrazione, ma anche del lavoro e dell'istruzione. un impegno complementare e coerente tra il Piano nazionale di ripresa e resilienza e la legge di delegazione europea per norme che attengono proprio alle stesse priorità strategiche, ovvero transizione ambientale verso un'economia verde sostenibile, con riferimento al VII programma quadro per l'ambiente e al *green new deal,* e transizione digitale, a cui molti articoli della legge di delegazione sono connessi. In questo quadro, di particolare rilievo sono gli articoli in materia di tutela del diritto d'autore e del mercato digitale, per mettere in relazione sviluppo delle tecnologie e tutela della creatività e del suo valore, anche in attesa di una disciplina europea che riesca a stabilire il giusto prelievo fiscale a carico di tali gestori, che operano in un mercato certo difficile da disciplinare, ma che è necessario regolamentare. Particolare attenzione ha posto il mio Gruppo all'articolo 3 per l'attuazione della direttiva 2018, che apre la strada a un contesto normativo più equo per il settore audiovisivo, verso una maggior tutela dei minori, per la lotta contro l'incitamento all'odio, nonché per prevedere misure nei confronti di chi utilizza profili fittizi al fine di alterare lo scambio di opinioni, generare allarmi e trarre vantaggio dalla divulgazione di false notizie. una tutela di estrema attualità, che ci appare necessaria non solo per i singoli, ma per la costruzione stessa del processo democratico. Di transizione ambientale si occupano poi molti articoli (5, 12, 19), in materia di mercato interno dell'energia da fonti rinnovabili, secondo il criterio della neutralità tecnologica, nonché secondo il principio del riuso e riciclo, verso un'economia compiutamente circolare; fonti rinnovabili e non inquinanti sia per l'autoconsumo che di comunità, con particolare attenzione al trasporto pubblico e, in prospettiva, anche a quello aereo in riferimento ai biocarburanti, nella consapevolezza che proprio la tutela della salute umana deve fare i conti con la salvaguardia dell'ambiente e il contrasto al cambiamento climatico. L'articolo 7 detta i princìpi in materia di pratiche commerciali sleali, nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare, e introduce elementi di maggior trasparenza a beneficio della stessa filiera dei consumatori finali. Se rendere più coese e convergenti le economie nazionali rende più competitiva l'economia europea, allora, signor Sottosegretario, è urgente sollecitare sui tavoli europei la riforma delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza, che ormai appaiono del tutto distoniche rispetto all'evoluzione di relazioni commerciali internazionali che richiedono una maggiore attenzione da rivolgere alle produzioni interne europee, ora che abbiamo compreso, anche a causa della pandemia, quanto la nostra economia debba contare sul mercato unico europeo. Per concludere, numerose sono ancora le procedure di infrazione a cui dare risposta, ben 83, con l'auspicio di accompagnare il lavoro di attuazione delle normative europee con un maggiore impegno in fase ascendente, ripensando anche a una più stretta collaborazione con le Regioni per le materie di loro competenza. Un lavoro, quello della partecipazione del nostro Paese alla costruzione europea, importante, che deve vederci protagonisti nell'interesse degli italiani e nell'interesse di un'Europa che venga percepita sempre più utile e vicina ai bisogni dei cittadini. Lo abbiamo detto, per questo serviva un Governo europeista; e oggi è il tempo di accelerare con coraggio. Ora la sfida è a casa nostra, per costruire e progettare oggi il futuro che lasceremo ai nostri figli, a partire dall'adozione di misure efficaci per contrastare la pandemia e tutelare la salute dei cittadini. Per questo torniamo a dire che non è più rinviabile l'utilizzo delle risorse del MES, ora che il sistema sanitario rischia di collassare di fronte al dilagare dei contagi. La sfida è di superare la crisi e di garantire ripresa e crescita durevole e strutturale, ma anche sostenibilità finanziaria delle misure adottate nel percorso verso la transizione verde e digitale. Anche la legge di delegazione contribuisce a tale trasformazione e a tale cambiamento. Per questo oggi noi facciamo la nostra parte, dichiarando il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-P.S.I. alla legge di delegazione europea 2019-2020.

anche quest'anno abbiamo il rito della legge europea; in sostanza, facciamo i compiti a casa. L'Europa ci dice quello che dobbiamo fare e noi lo facciamo. Ma lo facciamo ormai in modo talmente acritico che rischiamo di cadere veramente nel ridicolo. La relazione programmatica che ci accingiamo a votare è stata scritta a gennaio 2020, cioè prima della pandemia. La legge di delegazione europea ha cominciato il suo percorso anni fa, mesi fa, prima della pandemia, e noi facciamo finta che tutto questo non sia accaduto; facciamo i compiti a casa, facendo finta che il mondo sia lo stesso che c'era prima. Se voi credete di fare così la figura dei bravi europeisti, sbagliate; fate la figura degli imbecilli, perché uno deve essere anche minimamente razionale quando fa le cose. Fratelli d'Italia, nella sua proposta di risoluzione, chiede di ritirare i documenti e di ripresentarli adeguandoli al nuovo contesto, perché non facciamo una bella figura in Europa e non facciamo una bella figura in Italia. Dobbiamo dare seguito a 33 direttive, 14 regolamenti, 33 procedure di infrazione; ma, signor Sottosegretario, quante di queste saranno valide negli anni successivi? Vi sfugge che l'Europa ha deciso nuove regole, nuovi sistemi, nuovi aiuti alle imprese. Noi facciamo finta di nulla e andiamo avanti se nulla fosse. In ambito economico sono cambiate molte cose: i nuovi strumenti europei, la nuova funzione della BCE

dovevate essere più chiari e scrivere «gruppo» e, quando andavate in televisione, non dovevate dire che ci sono 800.000 euro a impresa, ma 800.000 euro di aiuti di Stato massimi per gruppo.

Sempre in ambito economico, Macron - che non mi sembra un sovranista - sta parlando di autosufficienza e di sussistenza. Banalmente dice: l'epidemia ci ha spiegato che una globalizzazione totale nella quale l'Europa non è autosufficiente quantomeno per la sopravvivenza è un problema. Macron domanda: ci poniamo il problema? Un

ragazzi, stiamo attenti; non è che domani non abbiamo neanche i prodotti alimentari di sopravvivenza? Non era il caso di parlarne nella legge di delegazione europea? No, parliamo dei 14 regolamenti che ci interessano e delle 33 direttive perché siamo in Europa in ginocchio da fermi e non capiamo qual è il ruolo della partecipazione dell'Italia in Europa. In ambito sanitario lo sapete che adesso stiamo andando verso il *lockdown*. La Francia e la Germania vanno verso il *lockdown*, ma ci siamo interrogati su una voce banale? all'applicazione di Schengen in periodo di pandemia. Quali sono le regole di ingaggio? Ognuno può chiudere all'altro, così come accaduto all'Italia quando vi siete fatti chiudere le frontiere in faccia da Francia, Slovenia e Austria perché eravamo gli appestati l'Europa? Adesso come funziona? Quali sono le regole? Era questa la sede per parlarne e non ne parlate perché il vostro documento è di gennaio del 2020.

cristiane ed europee. Per quanto riguarda lo Stato di diritto non spendete mai una sola parola in ordine alla questione del contrasto al fondamentalismo islamico in Europa. È un tema che Fratelli d'Italia affronta sistematicamente. In ambito europeo lo inserisce sistematicamente tra le priorità: lo abbiamo fatto negli anni scorsi e anche quest'anno,

avvengono episodi come quello di oggi, in cui terroristi islamici entrano dentro una cattedrale sgozzando e uccidendo delle persone. Qualche giorno fa era stato decapitato il professor Samuel Paty, colpevole di aver spiegato la laicità a scuola. È stato decapitato da un sedicente profugo ceceno, rifiutato dalla cristiana Polonia, finito in Francia a sgozzare ed ammazzare i professori francesi. Oggi abbiamo toccato il culmine della vergogna. Invito tutti a riascoltare gli interventi di dolore espressi dai

Nessuno di voi ha finora espresso solidarietà alla Francia e condannato l'omicidio islamista del professor Paty, perché credete che occorra assecondare qualunque forma di invasione dell'Europa e che parlare di integralismo islamico sia un tabù. *(Vivaci

è sintomatica la questione che dai banchi del PD arrivi l'urlo «fascista», perché sto dicendo che è una vergogna non condannare la decapitazione islamista del professore Samuel Paty, che non mi risulta essere un esponente di destra. Quindi, se il PD crede che condannare la decapitazione del professor Paty sia un atto da estremisti di destra siamo messi veramente male. Annuncio che, a differenza dei membri del PD, mi ha chiamato il sindaco dell'Aquila, l'amico Pierluigi Biondi, che ha annunciato che il Comune dell'Aquila dedicherà una via al professore Samuel Paty per ricordarsi esattamente quali sono le battaglie che dobbiamo compiere in Europa. e purtroppo ormai il MoVimento 5 Stelle con lui - che il ruolo dell'Italia in Europa sia quello di assecondare gli appetiti altrui: nessuna difesa dei nostri *asset* strategici, le nostre imprese saccheggiate questa debolezza arriva addirittura ad attaccare i nostri confini nazionali. Grazie a Fratelli d'Italia, abbiamo denunciato il tentativo di cedere parte delle nostre acque territoriali con l'accordo di Caen, che al momento è saltato; grazie a Fratelli d'Italia grazie a Fratelli d'Italia e all'interrogazione presentata dal senatore La Russa al Senato e dall'onorevole Lollobrigida alla Camera, abbiamo denunciato il tentativo francese di il tentativo francese di impossessarsi del vertice del Monte Bianco e anche questo speriamo che con la denuncia di Fratelli d'Italia sarà scongiurato Come ha recentemente detto il presidente del Partito dei conservatori europei, a nome dei 40 partiti europei occidentali che rappresenta, l'italiana Giorgia Meloni, non bisogna stare necessariamente in ginocchio davanti all'eurosistema, in Europa si può anche stare in piedi, a testa alta, a difendere il proprio interesse nazionale e il proprio popolo. È quello che intendiamo fare e per questo voteremo contro la pessima legge di delegazione europea di questo Governo.

un atto assolutamente fondamentale per il nostro Paese e particolarmente quest'anno, perché

legislativo, delle normative, è cruciale per il futuro dell'Europa. So che molte volte ci siamo trovati in situazioni

dell'occupazione. Pensiamo all'articolo 20 e ai principi e ai criteri direttivi specifici di delega per l'adeguamento al regolamento relativo al prodotto pensionistico, quello per i fondi per l'imprenditoria sociale, alla definizione di diritti minimi per i lavoratori e anche a quelli che riguardano l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare. Così come, nel campo della formazione e della cultura,

molto importante, che l'Europa ha come traguardo. Con questa legge di delegazione europea si interviene, per esempio, sulle energie rinnovabili, sapendo perfettamente che noi abbiamo discusso molte volte in questa Aula, sempre in vista dei Consigli europei, di quanto sia importante oggi, in questo momento, anche rispetto al programma Next generation EU, tutto il percorso verso la transizione energetica e i nuovi obiettivi che l'Europa che l'Europa si è data di riduzione delle emissioni, anche in vista del traguardo da conseguire della neutralità climatica nel 2050. Ci sono molti elementi che io trovo, dunque, non solo importanti, ma che ci mettono in grado anche di fare ulteriori passi in avanti.

ad alcuni emendamenti che, proprio sul fronte delle rinnovabili, sono stati approvati, a prima firma del collega Girotto, e che sono molto importanti per quanto ci riguarda. Noi li riteniamo

Per non parlare del fatto che abbiamo conseguito un obiettivo che ritengo abbastanza importante, anche rispetto

mi lasci dire, con cortesia,

Colleghe e colleghi, ci troviamo oggi ad approvare la legge di delegazione europea per gli anni 2019 e 2020. È stato un lavoro importante, che ha impegnato la Commissione per molte settimane, con l'esame dei testi, le audizioni, gli emendamenti. Un lavoro importante, e anche complesso, che ha visto il contributo di tutti i Gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposizione, che ringrazio insieme al mio predecessore, al Ministro, al sottosegretario Agea, a tutta la struttura della Commissione e ai relatori qui al mio fianco. Il disegno di legge può quindi passare alla Camera, sicuramente arricchito e migliorato, per la sua approvazione definitiva. Con la legge di delegazione approviamo anche le due relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per Intendo quindi procedere a sottolineare alcuni punti, perché credo sia opportuno farlo prima del voto. il rapporto con l'Europa. Il nostro Paese ha avuto in questi anni un rapporto con l'Europa contrastato, soprattutto per alcune posizioni critiche formulate nei confronti delle politiche della zona euro. Non tutte le posizioni critiche hanno evidenziato elementi di merito, ma alcune questioni le abbiamo poste anche noi, perché fondate. La costruzione europea, infatti, ha tuttora bisogno di un ammodernamento nelle sue istituzioni, nella sua *governance*, nelle sue regole di funzionamento. Ne siamo ben consapevoli. Ma è anche vero che i progressi maggiori sono stati realizzati nel corso dei periodi di crisi e ne abbiamo la riprova anche in questo tormentato 2020, in cui la pandemia da Covid ha provocato un grave *shock* economico, ma al contempo ha accelerato cambiamenti attesi da tempo. Faccio alcuni esempi. Si era parlato di regole di bilancio troppo stringenti, e il Patto di stabilità e crescita è stato sospeso; temporaneamente, ma è stato sospeso. Si era parlato di aiuti di Stato e di regole relative troppo rigide, e queste sono state sospese; anche queste temporaneamente, ma sospese. Si era parlato della BCE come troppo attenta al lato dell'inflazione, e abbiamo avuto la prosecuzione degli acquisti di titoli degli Stati membri. Si era parlato della necessità di dotare l'Unione europea di eurobond, e abbiamo avuto il meccanismo SURE e il *recovery fund*. Mi vengono in mente questi quattro aspetti per poter dire che si stanno facendo dei passi in avanti enormi nella costruzione della casa comune europea. Sono punti che ci fanno dire che una risposta europea c'è stata ed è stata molto forte. L'Europa non è il nemico che alcuni indicano in maniera quasi ossessiva, ma è la nostra grande opportunità, la nostra prospettiva di crescita, la nostra casa comune. Certo, Certo, questi aspetti andranno stabilizzati anche dopo la pandemia, quando sarà terminata, ed è questo l'orizzonte sul quale dobbiamo lavorare ed impegnarci. Non è infatti pensabile che gli avanzamenti che si sono realizzati e che hanno permesso di adottare politiche finalmente espansive siano solo temporanei. Ci dovrà essere tempo ed occasione affinché si apra una riflessione sulle modifiche definitive di alcuni paradigmi dell'Unione europea. D'altra parte, se anche il Governo federale tedesco ha previsto di aumentare il suo debito pubblico per 96 miliardi di euro nel 2021 per finanziare spese sociali e stimolare la ripresa economica, possiamo dire che qualcosa è davvero cambiato; ed è cambiato in meglio, anche grazie alla nostra azione. Resto all'oggi. In questi giorni abbiamo discusso molto e anche approfonditamente del *recovery fund*, anche qui in Aula. Si tratta della vera risposta europea alla pandemia ed è stato creato in uno spirito di solidarietà comune, che forse avremmo avuto difficoltà ad immaginare in tempi normali, anche recenti. Insieme con il meccanismo SURE, il *recovery fund* verrà finanziato tramite l'emissione di titoli obbligazionari da parte della Commissione europea: una svolta. Abbiamo chiesto per tanto tempo gli eurobond e ora abbiamo *bond* europei emessi dalla Commissione; ci si avvicinano molto e di questo dobbiamo esserne soddisfatti. Era una richiesta tutta italiana e ci siamo arrivati, per vie traverse, con una denominazione diversa, ma in qualche modo ci siamo arrivati. È un buon risultato del quale credo tutto il Parlamento dovrebbe gioire. Il secondo tema è il rapporto con gli Stati membri: la pandemia ha permesso di far comprendere a tutti che i nostri Paesi sono tra loro realmente interdipendenti. Non dobbiamo quindi in alcun modo esitare a riannodare i fili di un dialogo sempre più stretto con i nostri *partner* europei, per riuscire ad incidere maggiormente nella costruzione delle regole, cambiando paradigma. Non possiamo più dire che le direttive e i regolamenti ce li chiede l'Europa, perché l'Europa siamo noi, e non dobbiamo dimenticarlo. Partecipiamo anche noi ai negoziati e alle istituzioni che fissano le regole ed è lì che va esposto il nostro punto di vista, senza scadere nel lamento, ormai quasi rituale, che le regole europee si scrivono a Bruxelles, senza poi fare nulla per provare ad incidere nella loro definizione. Per fare questo, però, bisogna leggere i *dossier*, stabilire alleanze con gli altri Stati membri, ragionare in termini di famiglie politiche europee, dialogare con i nostri colleghi del Parlamento europeo. Certamente costa fatica e non porta molti consensi sui *social*, ma il nostro interesse nazionale lo tuteliamo a partire da questo *modus operandi*, cioè lavorando nella fase di costruzione della norma europea, per inserirci un pezzo più grande del nostro interesse nazionale, proprio come fanno gli altri Stati membri, anche perché non possiamo certo più dire che gli atti arrivano da Bruxelles senza che ce ne rendiamo conto: basti pensare alle direttive oggi contenute nel disegno di delegazione e che ci accingiamo a votare. Ognuna di esse è stata elaborata dal legislatore europeo, è vero, ma il nostro Senato, la Camera dei deputati e ogni altro Parlamento nazionale hanno la possibilità di esaminarle in tre momenti diversi: quando le proposte di direttiva vengono presentate a Bruxelles, quando esaminiamo il disegno di legge di delegazione europea e quando ci esprimiamo sugli atti del Governo che danno attuazione alla delega. Sono tre momenti distinti, che ci impongono di entrare nel merito delle singole questioni. Da questo punto di vista siamo assolutamente in grado di incidere sui contenuti della norma europea e di adattarli alle nostre specificità nazionali, ma bisogna lavorarci sopra, frequentare quei tavoli e motivare le nostre ragioni nei negoziati. In questo senso, come riferivo all'inizio del mio intervento, la legge di delegazione europea, oggi al nostro esame, contiene tante riforme importanti. C'è la delega per la riforma del sistema radiotelevisivo, che prendeva il nome del collega Gasparri; c'è quella per la riforma del sistema delle comunicazioni elettroniche, con il dibattito in corso sulla rete unica nazionale, dove si fissa il principio dell'accesso generalizzato alle reti di comunicazione ad altissima velocità e della loro diffusione, per tutti i cittadini, a prezzi accessibili; c'è la delega per la riforma del sistema di promozione dell'uso delle energie rinnovabili, che si innesta nel percorso di transizione verde, che sta compiendo c'è quella per la riforma delle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, che sono un nostro vanto nel commercio internazionale e che abbiamo il dovere di tutelare con forza. Sono solo i primi quattro articoli della legge di delegazione europea, che fanno però capire l'importanza cruciale di questo strumento normativo. Anche andando a verificare le direttive contenute nell'allegato, ci rendiamo conto dei temi decisivi che sono contenuti al loro interno. Prendo spunto dalle direttive in materia di giustizia:

Poi ci sono le direttive in materia di lavoro, come quella sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea e quella sull'equilibrio tra attività professionali e vita familiare. e vita familiare. In conclusione, cito l'approvazione dell'emendamento che introduce il divieto dei prodotti di plastica monouso, che impattano drammaticamente sull'ambiente, con cui cominciamo a rispondere in pieno alle missioni che ci siamo dati con il *recovery fund*. Sostenere al contempo la produzione degli stessi oggetti con plastica biodegradabile e compostabile e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile ha infatti un doppio rilevante vantaggio: facilitiamo la transizione *green*, dall'altra sosteniamo le nostre aziende che in questo settore sono all'avanguardia, perché è possibile mantenere e creare occupazione senza rinunciare all'ambiente e alla sua cura. Insomma, signor Presidente, la legge di delegazione europea permette al nostro Paese di adottare una serie di importanti riforme ogni anno, seguendo il modello sociale europeo cui ci siamo da tempo ispirati. Ecco perché il Partito Democratico, a nome del quale esprimo

Il loro approccio è stato costruttivo e non era per nulla scontato; anzi, devo dire che mi ha sorpreso perché in questi mesi ci siamo scontrati regolarmente con un atteggiamento di totale chiusura da parte del Governo e della maggioranza nei confronti delle nostre proposte, le quali ci avrebbero permesso di gestire in modo sicuramente più tempestivo e razionale l'emergenza sanitaria ed economica in corso. dopo aver dato il nostro via libera a scostamenti di bilancio per un ammontare complessivo di 100 miliardi di euro, siamo stati regolarmente esclusi da ogni tavolo di confronto e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: ritardi sopra ritardi accumulati nella gestione di una prevedibilissima seconda ondata di contagi; misure insufficienti a sostegno di imprese, partite IVA e lavoratori dipendenti; prestiti che si fa fatica anche solo a richiedere; risorse sperperate per l'acquisto di fantomatici banchi a rotelle e monopattini elettrici, responsabili - a mio parere - di uno scempio a danno delle nostre città in termini sia di decoro, che di sicurezza; mezzi pubblici pieni come uova. non ha ovviamente dato una risposta alla crisi e alla tensione sociale che purtroppo sta montando. Ci auguriamo, quindi, che il percorso positivo sperimentato in Commissione non rimanga un caso isolato, perché è inaccettabile che il Governo pretenda di gestire in totale autonomia i tanti, troppi, *dossier* sul tavolo. La collaborazione va praticata lo dico alla maggioranza - e non teorizzata, perché voi teorizzate la collaborazione, ma poi in pratica nessuna collaborazione c'è stata in questi mesi. In vista della complessiva sfida del Next generation EU, esigiamo dal Governo un coinvolgimento vero ai tavoli che decideranno il destino economico del nostro Paese e il futuro dei nostri figli. In ragione della situazione attuale, non dovrebbe essere più un tabù collaborare e lavorare insieme. Sia chiaro, non offriamo e non abbiamo mai offerto appoggio al Governo; solo ed esclusivamente la responsabilità e il senso delle istituzioni che oggi più che mai servono al Paese. di legge di delegazione europea in esame contiene la delega per il recepimento della direttiva sulla plastica, che prevede una serie di disposizioni che mirano a ridurne il consumo e trova un giusto bilanciamento tra la tutela dell'ambiente e la salvaguardia delle nostre realtà produttive. La direttiva indica la strada degli incentivi per sostenere la riconversione delle produzioni industriali: incentivi e non nuove tasse. Sia chiaro, le tasse non vanno aumentate, né trasferite, come invece vorrebbe fare il commissario Gentiloni con il gioco delle tre carte: dal lavoro alle cose, dal lavoro alla casa. La prima casa è un bene prezioso e non va toccata. Le tasse vanno diminuite; questa è l'unica strada per rilanciare l'economia e aiutare gli italiani stremati da questa emergenza che sembra non finire mai e che li sta portando alla disperazione. Nel testo è anche contenuta la delega per il recepimento della direttiva sul *copyright*. Si tratta di una direttiva importante cui hanno lavorato molto gli esponenti di Forza Italia anche al Parlamento europeo; la rete e i *social* sono un formidabile strumento di crescita, ma i giganti del *web* non possono continuare a saccheggiare le creazioni degli autori. *(Applausi).* Ho ritenuto doveroso quindi quindi sottolineare la questione del giusto compenso per giornalisti, scrittori, musicisti e artisti, presentando un ordine del giorno che è stato accolto dal Governo, che si è impegnato a definire per loro una remunerazione adeguata.

e migliorato la delega per l'attuazione del regolamento relativo al benessere degli animali, introducendo incentivi per chi sviluppa buone prassi di allevamento intensivo.

Non ci piace che la *governance* dei dispositivi medici sarà finanziata da chi dovrà controllare, cioè dalle imprese aggiudicatarie di gare d'appalto dei dispositivi medici stessi. Continuerò e continueremo quindi a lavorare perché questo evidente conflitto di interessi venga eliminato. Con la legge di delegazione europea votiamo oggi anche le relazioni del Governo sulla partecipazione del nostro Paese all'Unione europea. Su questo versante, colleghi della maggioranza e Governo, c'è veramente ancora molto da fare. Il Governo deve continuare a lavorare in Europa per un'equa armonizzazione fiscale, salvaguardando le nostre imprese dall'insopportabile fenomeno del *dumping* fiscale; Olanda, Lussemburgo e Irlanda fanno perdere all'Italia ben 8 miliardi di euro l'anno. Come denuncia il presidente dell'*Antitrust*, ogni anno sfuggono dalla tassazione del nostro Paese oltre 23 miliardi di dollari di profitti, che finiscono in giurisdizioni più favorevoli alle multinazionali. *(Brusio).* Prego anche i miei colleghi di Forza Italia di avere un minimo di

Non possiamo quindi più accettare che nell'Unione ci siano Stati che si comportano come veri e propri paradisi fiscali, attuando pratiche che danneggiano l'economia degli altri Paesi, compreso ovviamente il nostro.

In questo contesto mi sembra quindi anche doveroso sottolineare la necessità di un vero e proprio *reset* delle relazioni con la Cina: argomento scomodo, da mettere però necessariamente sul tavolo. Alla luce di ciò che sta accadendo nel mondo per responsabilità della Repubblica popolare cinese, non possiamo ancora fare finta di niente. Il rapporto dell'Italia e dell'Unione europea con Pechino non deve perdere di vista i nostri principi di riferimento. Dobbiamo pretendere dalla Cina il rispetto dei diritti umani, il rispetto delle regole a tutela dei lavoratori, anche a garanzia di una leale concorrenza economica, il rispetto della *privacy* a tutela della nostra sicurezza, il rispetto di norme igienico-sanitarie a salvaguardia di una comunità globalizzata e interconnessa, in cui le falle di un Paese si ripercuotono inevitabilmente su tutti gli altri. Il fatto che la Cina sia una potenza economica mondiale non può e non deve essere più un alibi a giustificazione del fatto che tutto le sia concesso. Serve un cambio di passo deciso e coraggioso da parte del nostro Paese e di tutta la comunità internazionale. Siamo molto preoccupati dalla deriva filocinese del Governo, come abbiamo detto più volte, e lo ribadisco in quest'Aula. i miei colleghi - a un gruppo cinese una parte consistente del porto di Taranto. Non possiamo continuare a piegarci a investimenti predatori da parte di Pechino. Voi avete un'enorme responsabilità nei confronti del futuro di questo Paese. Pechino, se vuole restare nel mercato globale, deve prima accettarne le regole. Serve il coraggio che non avete. Vi esortiamo a un cambio di passo e a farvi promotori, a livello comunitario, di iniziative volte a ottenere impegni precisi dalla Repubblica popolare cinese, a garanzia dell'economia e della salute di tutti noi. L'Italia, inoltre, deve ulteriormente lavorare affinché i nostri *partner* comprendano che le coste italiane corrispondono ai confini europei. Ci è stata presentata dalla Commissione europea una proposta di riforma del Regolamento di Dublino ma non mi sembra si sia compiuto alcun sostanziale passo in avanti. Ci attendiamo quindi che il Governo faccia sentire la sua voce affinché la riforma del regolamento di Dublino non sia solo uno *spot* ma venga fatta davvero. Se così non sarà, dopo la scellerata modifica dei decreti sicurezza e in particolare con il ripristino di quella che era una volta la protezione umanitaria, il nostro Paese sarà ancora più danneggiato da flussi che inevitabilmente si intensificheranno, alimentando le tensioni sociali che si susseguono

esigenze. Ci aspettiamo che prevediate dei ristori per queste famiglie e per queste aziende, che sono bloccate loro malgrado. Per tutti questi motivi dichiaro il nostro voto di astensione sulla legge di delegazione europea

le Relazioni programmatica e consuntiva annuali rappresentano lo strumento di controllo del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea. Questo documento, presentato dal ministro Amendola il 24 gennaio e annunciato in Assemblea il 18 febbraio di quest'anno, risulta anacronistico e quindi inadatto a descrivere gli impegni che l'Italia ha adottato e adotterà nell'Unione per l'anno corrente. L'emergenza pandemica da Covid-19, sorta in primavera, e la conseguente crisi economica mondiale hanno creato un prima e un dopo, come per le torri gemelle; tutto ciò che è stato scritto prima (valutazioni, prospettive e quant'altro) risulta oggi anacronistico, perché si rifà a uno scenario totalmente diverso. Oggi ci apprestiamo a votare con un atto di indirizzo una relazione che spiega gli impegni che l'Italia dovrà prendere in Europa per il 2020. Oggi è il 29 ottobre e l'anno termina il 31 dicembre. Come giustamente ha sottolineato il relatore, senatore Pittella, l'importanza di questo documento è nota a tutto il Parlamento. È questo il problema, la principale criticità: il Parlamento italiano, organo di rappresentanza del popolo italiano, tratta solo oggi, a sessantatré giorni dal 2021, le Relazioni programmatica e consuntiva e la legge di delegazione, continuando nei fatti ad essere completamente esautorato dal dibattito europeo. Cosa me lo fa pensare? Per esempio un Presidente del Consiglio che non permette il voto prima della sua partecipazione ai tavoli europei, sostenendo che sono informali, oppure il ritardo nell'invio di documenti importanti come abbiamo visto nella fase di trattativa di riforma del MES, ripeto, lo stesso dibattito di oggi completamente anacronistico e obsoleto. Nonostante l'assurdità della discussione in oggetto, approfitto per dire ciò che, secondo noi del Gruppo Lega-Salvini Premier, l'Italia dovrebbe fare in Europa. Mai come oggi è fondamentale ripensare ai parametri di Maastricht *(Applausi)*, prevedendo l'esclusione dal computo dei parametri utili al pareggio di bilancio e dal rapporto *deficit* - PIL degli investimenti produttivi, infrastrutturali, di messa in sicurezza del territorio, di quelli riguardanti la tematica ambientale e degli investimenti a favore della crescita demografica. Il tutto per permettere anche ai Paesi che devono perseguire la ristrutturazione del debito di poter rilanciare la propria economia investendo in settori strategici. Bisogna prevedere una reale semplificazione normativa per l'accesso ai progetti europei, considerando al contempo una revisione degli obblighi di cofinanziamento di fondi europei che spesso rappresentano un vincolo di spesa insostenibile in particolari realtà del Paese e che a volte comportano un mancato utilizzo di tali fondi. È necessario promuovere a livello europeo misure di valorizzazione delle eccellenze nazionali del *made in Italy* *(Applausi)* politiche coraggiose che proteggano le nostre imprese dagli attacchi predatori provenienti da Paesi dentro e fuori l'Europa. Questi sono tutti appelli che durante le audizioni i rappresentanti dei diversi settori del nostro tessuto produttivo ci hanno fermamente sollecitato. Queste sono preoccupazioni che si aggiungono a quelle che ci fanno temere per l'esistenza stessa dei nostri valori, della nostra storia e della nostra cultura, recentemente minata dalla scellerata ratifica della Convenzione di Faro. Non è questa l'Europa che vogliamo, un'Europa fatta di valori annacquati, o peggio negati, e prodotti surrogati: il cioccolato non cioccolato, il parmigiano non parmigiano o la dieta a base di insetti rispetto alla dieta mediterranea. È per questo che ci battiamo, per avere le risorse necessarie a difendere il nostro tessuto sociale ed economico. Questo è il motivo per cui riteniamo fondamentale assicurare, in sede di negoziato sulle proposte legislative per la nuova il mantenimento di adeguate risorse finanziarie o quantomeno analoghe al precedente quadro finanziario pluriennale dell'Unione, al fine di tutelare gli interessi nazionali e in grado di garantire un equo reddito ai produttori agricoli. difendere, in sede europea, il principio della sovranità e della tassazione diretta. L'attuale configurazione dell'Unione manca di sufficiente rappresentanza per imporre tasse a cittadini e imprese. Sul *green deal* europeo è evidente il diverso atteggiamento dell'Europa tra il settore produttivo della plastica, dove l'Italia è tra i *leader*, e quello del carbone che interessa particolarmente la Germania. Il processo di decarbonizzazione verrà sostenuto dai fondi europei. Il settore della plastica, probabilmente, sarà colpito da una nuova tassazione. L'unico risultato che questo comporterà sarà un calo di produzione della plastica in Europa, e quindi in Italia e se la pandemia continuerà si finirà per importarla da paesi extraeuropei che non rispettano alcun tipo di normativa. Tutto questo sicuramente non porterà alcun beneficio all'ambiente.

gli oli di palma e di soia per la produzione di biocarburanti. Sottolineiamo che questo, in primo luogo, contrasta con la direttiva europea, in secondo luogo rallenterà la conversione verso la mobilità sostenibile -, metterà in ginocchio le imprese della filiera della bioraffinazione che hanno investito centinaia di milioni. Bisogna evitare di assumere decisioni importanti in tema di neutralità climatica che incrementino gli obiettivi dell'Unione europea per il 2030 oltre il 40 Bisogna tener conto delle difficoltà economiche del momento e non si può permettere che i nostri agricoltori e le nostre aziende vengano vessate da tasse solo per ideologia. Si deve promuovere la nascita di un'agenzia europea per la cultura con sede in Italia, dal momento che il nostro Paese è primo al mondo per numero di siti dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO: sono 55 e dobbiamo valorizzarli con specifici progetti e investimenti, prevedendo una reale semplificazione normativa per l'accesso ai progetti europei. Dobbiamo ribadire la contrarietà dell'Italia riguardo all'adesione della Turchia all'Unione europea. *(Applausi)*. Questo alla luce delle sue azioni, che minacciano i nostri interessi energetici e strategici. Dobbiamo sostenere in ambito europeo la necessità di conservare un legame forte e privilegiato con gli Stati Uniti d'America e l'Alleanza atlantica; troppo spesso abbiamo sentito dichiarazioni ambigue da parte di esponenti di questa maggioranza e a volte del nostro Governo. Per quanto riguarda l'immigrazione, gli impegni dichiarati dal Governo per l'anno 2020 sono sconfessati nei fatti, con una gestione che ha consentito in questi mesi l'ingresso incontrollato di migliaia di immigrati irregolari che hanno messo a repentaglio la sicurezza sanitaria dei nostri cittadini. Invitiamo il Governo ad assumere tutte le iniziative ritenute utili per promuovere un rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione europea, al fine di contrastare la tratta degli uomini e la criminalità organizzata a essa connessa. L'Italia deve impegnarsi al fine di disincentivare le partenze e sostenere la creazione, nei Paesi di partenza e transito, di appositi centri in cui avviare gli immigrati per verificare da subito la sussistenza dei requisiti richiesti per l'asilo politico.

Non si sa quali siano le condizioni, perché sui mercati i tassi sono negativi. Quanto ci costano i tassi dell'Europa è vietato saperlo, perché è stato tutto segretato. È questa la trasparenza? Dal momento che abbiamo il sentore, anzi la quasi certezza che questo Governo non sarà in grado di garantire quelle che per noi le priorità per l'Italia in Europa, con il presente comunico il voto contrario della Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione su tutti e due i documenti in esame.

finalmente arriviamo alle battute finali, dopo un lunghissimo e travagliato percorso prima in Commissione e poi anche in Aula. Non ricordo che una legge di delegazione abbia mai preso tutto questo tempo. di vedere, è stato anche appesantito da interventi spesso fuori luogo e inopportuni, fatti dal principe degli assenteisti in Senato, che vediamo solo in determinate occasioni e per usare questa Aula come palcoscenico per attaccare il Presidente del consiglio e il Governo. *(Applausi)*. Stiamo trattando di legge di delegazione europea e invece ho visto tantissimi interventi anche sugli emendamenti; ognuno si sente libero di intervenire sulla legge delegazione europea per trattare il tema che reputa più opportuno e utile anche a fomentare l'odio religioso e razziale. Dovremmo restituire a quest'Aula la necessaria dignità. Perciò anch'io divago ed esco fuori dal seminato della legge europea... Signor Presidente, qui c'è qualcuno che, appena viene additato dai colleghi, si alza dicendo che gli impediscono di parlare. Io mi rivolgo a lei, signor Presidente, e chiedo che i colleghi abbiano rispetto, come lo abbiamo noi dall'inizio alla fine.

Torniamo ai temi della legge di delegazione europea. Ringrazio il relatore, i presidenti e il sottosegretario Agea perché hanno avuto anche loro tanta pazienza, però mi permetto di invitare

consentite all'Assemblea e alle Commissioni di lavorare per bene perché i temi delle direttive europee e dell'Europa tutta per noi sono importanti. Perciò, mi permetto di fare un invito al Governo e al Ministro Nello specifico la legge interviene, ad esempio, sulla disciplina dei servizi dei *media* audiovisivi, delegando al Governo un riordino generale della normativa recependo, altresì, cambiamenti intervenuti in Europa in materia di tutela della dignità umana e dei minori,

Si interviene ancora in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola, al fine di tutelare meglio i produttori (e l'attenzione di questa maggioranza e del Governo per i produttori agricoli è sempre molto alta). I temi sono molti e perciò cerco di evitare un mero elenco. Vorrei solamente soffermarmi su alcune questioni che ritengo maggiormente significative.

un tema fondante. Grazie a questa norma ci avviciniamo a grandi passi all'idea di futuro che abbiamo in mente da undici anni: energia pulita da fonti rinnovabili del cittadino e a servizio dello stesso. Vorrei citare le comunità energetiche, anche questo è un tema a noi molto caro, già anticipate nel milleproroghe del 2020 e da un decreto del Ministero dello sviluppo economico di poche settimane fa. In merito, ringrazio anche Stefano Patuanelli per l'impegno profuso. compiamo un ulteriore passo in avanti verso la creazione di un quadro giuridico semplice e omogeneo in grado di contribuire alla loro necessaria espansione. Per noi le comunità energetiche sono importanti per superare anche la dipendenza dalle fonti fossili e perciò anche da fonti esterne alla Nazione, un altro punto del programma del Movimento che viene realizzato sempre con l'intento di mettere il cittadino al centro e fornirgli gli strumenti per essere parte del cambiamento verso un futuro non più rimandabile, grazie anche alle risorse del *recovery fund* per cui il Presidente del Consiglio si è battuto e che ringrazio per questo. Abbiamo un'occasione unica per realizzare quanto detto. Recepiamo, inoltre, il codice delle comunicazioni elettroniche, che costituisce anche in questo caso un nuovo passo verso l'ammodernamento del nostro Paese. Paese. Seppure la rete italiana abbia superato la prova del *lockdown* - ricordiamo che nei giorni di chiusura totale non era scontato

che alcune zone del Paese vivono quotidianamente. Pensiamo alle difficoltà incontrate da alcuni cittadini a causa dell'assenza di una connessione adeguata allo svolgimento dello *smart working* o della didattica a distanza. Bene, con questo provvedimento si pongono le basi per il rinnovamento della rete e per un suo sostanziale potenziamento mirante, tra l'altro, al superamento della condizione di esclusione delle zone bianche ancora presenti nel Paese per cui si è intervenuti in Commissione. Altro tema fondante affrontato da questo disegno di legge è quello ambientale. Penso immediatamente

La prima mira a limitare l'utilizzo dei prodotti in plastica monouso al fine di prevenirne la dispersione nell'ambiente e nel mare, mentre la seconda mira a dotare i porti di impianti di conferimento dei rifiuti adeguati e che rispettino i principi dell'economia circolare. Credo sia evidente anche ai più distratti come l'azione del Governo, anche in questo caso, anticipi il recepimento della normativa europea e ne apra la strada: penso al disegno di legge cosiddetto salvamare, che ha visto riprendere il suo *iter* proprio qui in Senato dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia; alla *plastic tax* e agli interventi per il rinnovamento del parco auto circolante per la transizione verso la mobilità elettrica, che stiamo incentivando da prima dello scoppio della pandemia globale. soprattutto a quanto approvato il 13 ottobre scorso qui in Senato in relazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'ambiente è al centro dell'azione di Governo e della maggioranza

Proprio in tema di SUP credo sia importante anche sottolineare come, grazie all'intensa attività di mediazione tra Parlamento e Governo, sia stato approvato un emendamento di grande importanza, non solo per l'ambiente ma anche per l'Italia: mi riferisco alle bioplastiche, quelle biodegradabili e compostabili, quali sostituto della plastica quei contenitori monouso per cui non sia possibile avere un'alternativa riutilizzabile. L'approvazione di questo emendamento non solo tutela l'ambiente, ma dà sicurezza a una filiera che ci vede *leader* in Europa e che rischiava di venire danneggiata da una non corretta interpretazione delle norme comunitarie. Vorrei citare un ulteriore emendamento volto a chiarire un'ambiguità che si era creata in relazione alla possibile esclusione dei bicchieri di plastica monouso dalla normativa. Grazie a questo emendamento, fortemente voluto dal MoVimento 5 Stelle e da tutta la maggioranza, superiamo i rischi di un non corretto recepimento della direttiva e creiamo un ambiente favorevole per le nostre aziende italiane che potranno godere di un quadro normativo certo per poter pianificare la transizione verso un mondo libero dalla plastica monouso. Tutto questo per dire che, seppure la pandemia ha sicuramente rallentato i lavori che hanno portato questo disegno di legge in Aula, il testo che oggi è sottoposto all'esame è il frutto di un grande impegno e di una sinergia creata tra Governo, Parlamento e opposizioni e rispecchia la visione che abbiamo del Paese per i prossimi anni. La ripartenza è stata ed è complicata... Ma oggi diamo alle imprese e a tutti gli altri attori un quadro normativo maggiormente chiaro e omogeneo che gioverà alla ripresa delle normali attività economiche e allo sviluppo dell'Italia. Per questi motivi e per tutto quello che abbiamo fatto finora e che faremo esprimo il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

L'ordine del giorno reca: «Informativa del Presidente del Consiglio dei Ministri sul DPCM del 24 ottobre 2020, recante ulteriori misure per il contrasto della diffusione dell'epidemia da COVID-19». Ricordo che è in corso la diretta televisiva con la RAI.

Signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, torno qui, in Parlamento, per illustrare le ulteriori misure restrittive,

Come è noto, nella sera di sabato 24 ottobre ho firmato un nuovo decreto, all'esito di un lungo e articolato confronto tra tutte le forze di maggioranza, con i Presidenti di Regione e con il Comitato tecnico-scientifico. Nel pomeriggio di sabato ho inoltre, doverosamente, informato i Presidenti delle Camere della mia intenzione di venire a riferire, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 19 del 2020, sul contenuto delle ulteriori misure adottate. D'accordo con i Presidenti dei due rami del Parlamento, ho poi voluto informare i Presidenti dei Gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione sulle importanti determinazioni che stavamo per assumere e li ho incontrati lo stesso pomeriggio di sabato 24. I dati delle ultime settimane indicano una curva epidemiologica in rapida crescita, con diffusione del virus su tutto il territorio nazionale. L'indice RT ha raggiunto la soglia critica di 1,5 e il numero di nuovi positivi al virus è cresciuto in maniera preoccupante. Risulta ormai difficoltoso per gli operatori tracciare in modo completo le catene di trasmissione. Lo stesso, peraltro, sta avvenendo in molti altri Paesi europei, in particolare in Germania e Francia, come ammesso pubblicamente rispettivamente dalla cancelliera Merkel e dal presidente Macron. Questo quadro epidemiologico sta determinando una pressione particolarmente severa sul nostro servizio sanitario. Negli ultimi giorni si è infatti osservato un incremento significativo del numero di persone ricoverate e conseguentemente sono aumentati i tassi di occupazione delle degenze in area medica e in terapia intensiva. Da tutto ciò deriva la necessità di adottare misure che consentano di raffreddare e mitigare il più possibile la curva di crescita del contagio, al fine di alleviare il carico già molto pesante che grava sul sistema sanitario. Riassumo di seguito le ragioni e anche i criteri che hanno ispirato queste ultime scelte. Innanzitutto, mi preme sottolineare che le misure adottate

tutte sempre ispirate ai principi di massima precauzione, adeguatezza e proporzionalità e mai tendenti a sottovalutare la severità e l'imprevedibilità della pandemia. Non abbiamo mai affermato di essere fuori dal pericolo e da una costante condizione di necessaria allerta. In questi mesi abbiamo agito di conseguenza, impegnandoci costantemente nell'attuazione di una pluralità di misure atte a realizzare un adeguato apparato di prevenzione del contagio e di rafforzamento del servizio sanitario. Notevole è stato lo sforzo sin qui compiuto in termini sia finanziari che organizzativi per potenziare l'organizzazione del servizio sanitario. Tali interventi appaiono tanto più rilevanti se si ha la bontà di considerare che negli ultimi anni il reiterarsi delle diverse misure di contenimento della spesa aveva determinato una significativa riduzione anche del personale del Servizio sanitario nazionale. Nella prospettiva di consolidare e stabilizzare l'apparato preventivo costruito e nella consapevolezza di non aver superato la fase del rischio pandemico si iscrive la scelta

e successivamente a ottobre, quando invece già si palesava una nuova recrudescenza del contagio. Ricordo che tale decisione, da parte di alcuni (anche tra i presenti in quest'Aula) fortemente criticata, ha in realtà consentito di mantenere in vigore quel quadro giuridico che costituisce il presupposto per l'intera nostra disciplina dell'emergenza, nonché per la continuità operativa del sistema di allerta, prevenzione e contrasto del virus. Le misure si collocano pertanto in un *continuum* di interventi progressivamente più restrittivi e rigorosi, adeguati all'evoluzione dell'epidemia che si muove con crescente e preoccupante rapidità. Con le misure adottate da ultimo lo scorso 24 ottobre abbiamo compiuto il passo più deciso; abbiamo scelto di intervenire su attività, ambiti e situazioni suscettibili di favorire direttamente o anche indirettamente fenomeni aggregativi e afflussi eccessivi di persone, spesso concentrati in determinati orari della giornata. Le misure introdotte si fondano sulle indicazioni e le raccomandazioni elaborate dai nostri esperti e scienziati e fanno riferimento anche a protocolli internazionali formulati per il contrasto alla pandemia. Vorrei sottolineare in particolare che l'Istituto superiore di sanità, insieme e d'intesa con il Ministero della salute, la Conferenza delle Regioni e vari organismi di ricerca anche universitari, hanno pubblicato, ed è quindi accessibile a tutti, il documento che vi invito a considerare intitolato «Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione autunno-invernale». In questo documento sono rappresentate, in relazione all'evoluzione di scenari epidemiologici, le specifiche e diverse modulazioni delle misure da adottare. Allo stato l'epidemia è in rapido peggioramento e risulta compatibile a livello nazionale con lo scenario di tipo 3, che è descritto nello studio, con rapidità di progressione maggiore in alcune Regioni italiane. In particolare, per lo scenario di tipo 3, lo studio menzionato prevede tra le misure da adottare proprio quelle alle quali il Governo si è attenuto. Non abbiamo quindi agito secondo criteri arbitrari, né operando una impropria gerarchia di valori tra differenti attività con il risultato di apprezzarne alcune a scapito di altre, ma ci siamo attenuti a evidenze scientifiche che ci hanno consentito di compiere solide valutazioni prognostiche. Non solo,

Con verbale n. 121, reso qualche ora più tardi dello stesso giorno, il CTS - leggo letteralmente - «dopo ampia analisi condivide i provvedimenti previsti dal testo». poi aggiunto qualche limitata osservazione che peraltro il Governo ha sostanzialmente recepito. Voi sapete che il regime di pubblicità degli atti del CTS prevede la pubblicazione, quindi l'accessibilità a tutti, dopo il verbale n. 121 sarà pertanto accessibile integralmente tra un po' di giorni. Peraltro, la *ratio* che ha ispirato le misure è coerente con il modello adottato per la fase di ripresa delle attività. quindi una coerenza nella strategia del Governo per affrontare e gestire la pandemia. Infatti il nostro modello, che ha portato alla creazione di quattro classi di rischio - basso, medio-basso, medio-alto e alto - è basato su tre parametri: esposizione, prossimità e aggregazione. Come è noto, la riapertura progressiva delle attività ha interessato prima alcune classi di attività lavorative, poi quelle commerciali e, infine, quelle che potremmo definire ludico-ricreative. Per questo, nel momento in cui siamo costretti a progressive restrizioni, quindi adesso, dobbiamo inevitabilmente adottare i medesimi criteri, procedendo però a ritroso, a partire da quelle attività che presuppongono e determinano propensione alle relazioni sociali anche, se non soprattutto, tra persone sconosciute. In particolare l'intervento si è decisamente indirizzato con maggiore severità a tre settori: ristorazione serale, teatri, cinema e sale concerto, palestre e piscine, le cui attività sono state sospese. Sono, inoltre, sospese tutte le competizioni sportive, ad eccezione di quelle professionistiche a livello nazionale, senza, però, più la presenza del pubblico. Per ciò che concerne l'attività sportiva di base, rimane consentita solo quella non da contatto e comunque al di fuori di palestre e piscine. Entro la medesima logica si iscrive l'estensione del divieto di organizzare feste, anche con riferimento a festeggiamenti conseguenti a cerimonie civili o religiose, del Consiglio dei ministri del 13 ottobre potevano essere svolte nel limite massimo di 30 persone. Così come si iscrive in questa medesima logica

Ugualmente ispirata a una logica di contenimento delle occasioni di aggregazione e di incontro è la raccomandazione di non spostarsi, salvo che per esigenze lavorative, di studio, di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Questo complesso apparato di divieti, sospensioni, raccomandazioni è stato oggetto di critiche, anche molto accese, da parte innanzitutto delle categorie direttamente interessate, ma anche da parte di molti cittadini, che hanno espresso il loro dissenso, anche con manifestazioni di protesta spontanee in alcune città. Ai soggetti coinvolti tali scelte sono apparse in contraddizione con l'obbligo di adottare rigorosi protocolli di sicurezza, che è stato, come ricorderete, uno dei presupposti che ci ha consentito, a partire dal mese di maggio, la progressiva riapertura delle medesime attività. Sul punto, tuttavia, desidero ribadire ancora una volta che la scelta di sospendere o ridurre temporaneamente l'attività in alcuni settori qui, come in altri Paesi europei - non deriva dal mancato rispetto delle misure di sicurezza che, salvo eccezioni, sono state adottate anche con rigore e a prezzo di sacrifici e di non trascurabili costi di organizzazione. Se siamo stati costretti a operare scelte così radicali, la causa risiede esclusivamente nell'esigenza di ridurre, in presenza di un contagio diffuso ed esponenziale, senza che possano identificarsi precisi, circoscrivibili focolai, focolai, le occasioni di socialità, di relazione, soprattutto in quei contesti in cui è più facile che venga abbassata la guardia e quindi vengano allentate le indispensabili precauzioni del distanziamento e dell'uso dei dispositivi di protezione personale. Inoltre, oggettiva difficoltà - di assicurare sempre il rigoroso rispetto delle regole di distanziamento sui mezzi di trasporto, anche nelle ore di maggiore afflusso degli utenti, unita al mancato pieno utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Governo da parte delle Regioni per servizi aggiuntivi di trasporto locale (risultano al momento utilizzati 120 milioni di euro dei 300 messi a disposizione), impone di alleggerire la pressione sul trasporto pubblico e privato, limitandolo solo agli spostamenti di necessità, evitando per quanto possibile assembramenti alle fermate o all'interno dei mezzi. Ribadisco che, a differenza di quello che viene imputato al Governo, le attività che sono state sospese non sono state sospese perché ritenute non essenziali; si tratta di attività pur sempre fondamentali - e il Governo ne è pienamente consapevole - per il benessere della persona che, anche sulla base di ormai consolidate acquisizioni mediche, presuppone la cura del corpo, ma anche il nutrimento dello spirito. La scelta discende esclusivamente dalla necessità, fondata su evidenze scientifiche, di diradare il più possibile i contatti sociali e le interazioni tra le persone.

Anche questa misura ci è costata molto, soprattutto considerando l'intenso lavoro svolto nei mesi estivi per dotare la scuola di un sistema di prevenzione e di sicurezza tale

Analogamente, risponde alla medesima *ratio* l'incentivazione nelle pubbliche amministrazioni allo *smart working* e alla differenziazione dell'orario di ingresso del personale. Questa modalità di lavoro, peraltro, è raccomandata anche nel settore privato. Permettetemi di soffermarmi, in particolare, sulla misura con la quale abbiamo sospeso gli spettacoli nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche. Ho già avuto modo di affermarlo in più sedi: questa scelta è stata particolarmente dolorosa. I protagonisti del mondo dello spettacolo, parlo degli artisti, musicisti, autori, imprenditori, tecnici e lavoratori stanno affrontando ormai da molti mesi enormi difficoltà che aggravano una condizione che possiamo definire di criticità strutturale, viste ormai le nuove tecnologie che rischiano di oscurare la magia che scaturisce dalla tradizionale fruizione di concerti e rappresentazioni teatrali e cinematografiche nelle sale aperte al pubblico. Purtroppo, gli stessi protocolli di sicurezza, seppure hanno offerto garanzie per evitare il contagio nelle sale, tuttavia negli scorsi mesi hanno fortemente limitato la presenza del pubblico, contribuendo a un generale depauperamento dell'intero settore. Peraltro, siamo consapevoli che il danno recato a questo settore deriva anche dalle modalità di organizzazione che si basano su una programmazione non di breve periodo. Questo significa che, da un lato, la chiusura interrompe attività sulle quali si era investito sotto il profilo delle risorse umane e finanziarie già da tempo, quindi chiude la prospettiva di ricavi che erano stati ovviamente frutto di investimento; dall'altro, la medesima riapertura delle attività, che speriamo avvenga il prima possibile, non significherà immediata ripartenza proprio considerata l'esigenza di una adeguata programmazione. Questa scelta ci pesa anche, se non di più, per il significato che la chiusura di questi luoghi implica, per il loro valore sociale e culturale, non solo economico. Sappiamo quanto in quegli spazi - parlo, appunto, dei teatri, dei cinema e delle sale da concerto - la persona nutra lo spirito e articoli la capacità di definire la propria identità, finanche la propria emotività. In quei luoghi si rafforza il sentimento di appartenenza ad una dimensione collettiva, si cementa la medesima coesione sociale che si alimenta della condivisione di quei valori di civiltà tanto più essenziali in un momento così duro di crisi come quello che l'umanità sta attraversando. Il Governo è pienamente consapevole degli immani sacrifici richiesti a tutte queste categorie di lavoratori e da subito si è posto in ascolto. Siamo estremamente sensibili alle manifestazioni di dissenso, protesta e frustrazione che si sono verificate in questi giorni in alcune città d'Italia: cittadini e lavoratori che esprimono pacificamente il proprio disagio, le proprie angosce e paure, che vedono minata la propria sicurezza economica e temono per il futuro delle proprie attività e del proprio lavoro. È per questo che abbiamo ritenuto giusto confrontarci immediatamente con i rappresentanti delle categorie più penalizzate dalle nuove misure restrittive al fine di spiegare loro direttamente le ragioni sottese a questi interventi e di annunciare le proposte di ristoro e di indennizzo individuate tempestivamente dal Governo. Consapevoli fin dall'inizio dell'impatto che queste restrizioni avrebbero avuto su un gran numero di attività commerciali, produttive, culturali e sportive e sui lavoratori impegnati in questi settori, il Governo ha infatti parallelamente - nelle medesime ore in cui lavoravamo per le misure restrittive - predisposto adeguati strumenti di intervento a supporto di tali categorie,

squilibri preesistenti e generando nuove diseguaglianze. Rivendico questa come una decisa e qualificante scelta di politica economica e sociale.

che forniscono un sostegno immediato, consistente e aggiuntivo rispetto a quello predisposto all'inizio della pandemia e nei mesi scorsi. Il pacchetto di misure previste dal decreto-legge è complessivamente quantificabile in 5,4 miliardi di euro, se parliamo di indebitamento netto, e in 6,2 miliardi in termini di saldo netto da finanziare. Innanzitutto, oltre 2 miliardi sono stati riservati a un nuovo contributo a fondo perduto per le attività dei comparti interessati dalle nuove disposizioni, con livelli di ristoro e di indennizzo differenziati a seconda dell'intensità del danno economico subito dalle categorie. Abbiamo individuato quattro fasce, con diverse scale di coefficienti di ristoro (100, 150, 200, fino a 400 per cento), con riferimento alle compensazioni già ricevute secondo quanto previsto dal decreto-legge rilancio. Per quanto riguarda le modalità di erogazione, è previsto un doppio binario: coloro che in precedenza avevano presentato la domanda per la prima edizione del contributo a fondo perduto riceveranno, entro la metà di novembre, un bonifico da parte dell'Agenzia delle entrate direttamente sul conto corrente che il beneficiario ha già indicato.

fondo perduto, in quanto avevano un fatturato superiore ai 5 milioni di euro, adesso invece potranno presentare richiesta e il ristoro sarà corrisposto in modalità identiche - confidiamo già per la metà di dicembre - con una nuova procedura avviata verso la metà di novembre. In aggiunta, per ulteriori sei settimane saranno rifinanziate la cassa integrazione ordinaria (l'assegno ordinario) e la cassa integrazione in deroga legata all'emergenza Covid-19. Contestualmente sarà riproposto il reddito di emergenza, con due nuove *tranche* mensili a partire da 400 euro esigibili da tutti coloro che ne avevano già diritto e da chi nel mese di settembre ha percepito un reddito familiare inferiore al beneficio stesso. A favore delle filiere dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura è stato istituito un fondo da 100 milioni di euro, volto a concedere contributi a fondo perduto alle imprese del settore. Abbiamo inoltre stanziato un miliardo di euro a sostegno del mondo della cultura e del turismo, mentre significative risorse sono state stanziate in favore dei lavoratori del settore sportivo e delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Abbiamo predisposto infine un insieme di interventi volti a rafforzare la risposta sanitaria all'emergenza epidemiologica. Tra questi segnalo in particolare 30 milioni di euro per favorire la somministrazione di tamponi rapidi presso i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. È proprio di ieri il fatto favore - che sono stati sottoscritti due nuovi accordi collettivi, rispettivamente per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta, che contemplano tra le nuove clausole clausole la possibilità di coinvolgere queste categorie professionali e di operatori sanitari nell'attività di rafforzamento dell'opera di prevenzione e prevedono il coinvolgimento di questi medici nell'attività di indagine epidemiologica e anche per i test. È un fatto molto importante perché alleggerisce molto l'intensa attività e il sovraccarico in questo momento del dipartimento di prevenzione. Occorre sottolineare che l'impegno del Governo italiano per il superamento della crisi da Covid si dispiega, fin dall'inizio della pandemia, anche in sede europea e multilaterale. Senza una risposta coordinata a livello dell'Unione europea e sul piano globale, nessuno Stato può da solo superare la crisi sul piano sia sanitario che economico. L'attenzione dell'Unione europea rimane alta, tanto più a seguito della recrudescenza del Covid nel nostro continente in queste ultime settimane. Questa impostazione abbiamo messo a punto in particolare anche nell'ultimo Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. Leggo testualmente dalle conclusioni di quel Consiglio europeo: «Ha invitato il Consiglio stesso, la Commissione e gli Stati membri a proseguire lo sforzo globale di coordinamento sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, in particolare per quanto riguarda le norme di quarantena, il tracciamento transfrontaliero dei contatti, le strategie in materia di test, la valutazione congiunta dei metodi diagnostici, il riconoscimento reciproco tra gli Stati dei test, la limitazione temporanea dei viaggi non essenziali europea». Il medesimo Consiglio: «ha ribadito la necessità di definire un solido processo di autorizzazione e di monitoraggio, creare capacità di vaccinazione nell'Unione europea garantire un accesso ai vaccini equo e a prezzi abbordabili» e «i *leader* hanno incoraggiato la cooperazione a livello mondiale». In sostanza, la competenza in materia di salute rimane certamente nazionale, ma i capi di Stato e di Governo degli Stati membri, gli stessi vertici delle istituzioni comunitarie hanno concordato sulla necessità di un coordinamento efficace perché ci renderà tutti più forti. Potremo prevenire meglio e superare le criticità sul piano sanitario. In quest'ottica di condivisione e di coordinamento europeo, proprio questo pomeriggio - tra poco - si farà un punto sulla situazione sanitaria. Ci sarà una videoconferenza con tutti i *leader* europei e i vertici delle istituzioni comunitarie.

che l'Esecutivo comunitario ha adottato mercoledì 28 ottobre e che mira appunto a favorire un adeguato coordinamento continentale sul piano sanitario, in particolare sulle strategie di test e sul vaccino anticovid. Alla videoconferenza di questo pomeriggio ne seguiranno altre perché nell'ultimo Consiglio europeo abbiamo concordato di scambiare informazioni e confrontarci costantemente in modo da proseguire uniti, per quanto possibile, nella strategia di contrasto della pandemia. Io stesso ho suggerito, proprio nell'ultimo Consiglio europeo, di affiancare ai *leader* anche i Ministri della salute, i quali sono impegnati in prima linea sul piano tecnico. Quindi, questo pomeriggio avrò a fianco

una positiva conclusione del negoziato su Next generation EU e sul nuovo quadro finanziario pluriennale, perché far partire al più presto i programmi e l'erogazione dei fondi europei rappresenta innanzitutto un obbligo morale verso le decine di migliaia di vittime europee e verso i cittadini del nostro continente. L'Italia resta impegnata a tal fine in una serrata e intensa azione politico-diplomatica a tutto campo. Mi avvio alla conclusione. Il rinnovato impeto del virus ci pone di fronte a una nuova sfida, non meno minacciosa della prima battaglia che abbiamo combattuto la scorsa primavera. È una seconda sfida che continua a investire tutto il mondo e con una cresciuta intensità - come possiamo tutti constatare - tutta l'Unione europea.

Ormai un po' tutti i Paesi europei hanno introdotto misure restrittive, in alcuni casi anche più severe delle nostre, per proteggere la salute dei cittadini e le proprie economie. Tutti i Governi europei, con i loro meriti e i loro demeriti - questo vale ovviamente anche per questo Governo - stanno fronteggiando un nemico che oggi ci costringe a fare un passo indietro. Siamo quindi costretti a modificare alcune abitudini di vita e i nostri comportamenti. La scorsa settimana il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ci ha ricordato che tutte le articolazioni dell'ordinamento democratico, per perseguire il benessere della società e lo sviluppo dei territori, sanno di dover operare sempre con spirito di unità e di coesione, consapevoli dei tanti interessi comuni. Questo è il momento di restare veramente uniti.

Dobbiamo restare uniti, pur nella varietà delle opinioni, pur nel rispetto delle differenti sensibilità. Ringrazio coloro che hanno sostenuto i nostri sforzi protesi a salvare tanto le vite umane, quanto il tessuto produttivo del Paese, e tutti coloro che, pur nella legittima dialettica politica che caratterizza e deve caratterizzare una moderna democrazia, offrono un contributo costruttivo ai nostri sforzi protesi al bene e all'interesse del Paese. Regnano ancora una grande incertezza e insicurezza sulla fase che stiamo attraversando. Vi assicuro che il Governo ce la metterà tutta per mettere in sicurezza il Paese. Tutti noi componenti del Governo siamo consapevoli che dobbiamo impegnarci con tutte le nostre energie e tutta la nostra determinazione in questo compito. In particolare, siamo pienamente consapevoli che siamo qui non per noi, «siamo qui per gli altri uomini: innanzitutto per coloro dal cui sorriso e dal cui benessere dipende la nostra felicità, ma anche per quella moltitudine di sconosciuti alla cui sorte ci incatena un vincolo di simpatia».

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi,

stiamo vivendo un tempo decisamente diverso da quello che l'Italia ha vissuto nella primavera scorsa: è il tempo che si è aperto in questo autunno e - bisogna riconoscerlo - è decisamente peggiore. Dovremmo fare ammenda - non soltanto chi è qui, ma anche chi è fuori da qui - per aver dimenticato nel periodo estivo che dopo l'estate veniva l'autunno e che abbassare la guardia fuori da qui e dentro le Aule parlamentari si sarebbe rivelato un tragico errore. Io non appartengo alla categoria di chi soffia sul fuoco, ma trovo altrettanto colpevole sia chi soffia sul fuoco, sia chi eleva il silenzio a motivo, a ragione, a comportamento. Questo non è il tempo per manifestare in un'Aula parlamentare Quello che abbiamo fatto in passato lo rifaremo e lo rifarò e cioè consegnare la fiducia di un Gruppo, di una storia politica e di una persona che parla in quest'Aula e parla a lei, decisamente nelle sue mani. Prima che essere partigiani di una parte e partigiani di un'idea, siamo italiani e tali siamo fuori e dentro quest'Aula. Mi consenta, però, tre considerazioni che riguardano l'Assemblea, ma che riguardano in modo particolare il Governo. Lei ha inneggiato continuamente al confronto: condivido, sottolineo e sottoscrivo. Quando si entra in un'Aula parlamentare,

continuo a sostenere che, da questa seconda fase molto più delicata della prima, si esce solo se si genera, solo se germina dall'attività parlamentare e dall'attività del Governo un nuovo spirito civico, ed è il secondo punto che affronto. Lei ha pronunciato, alla fine del suo intervento, un appello a restare uniti. Sottoscrivo anche questo, presidente Conte, ma non basta l'appello a restare uniti. uno spirito civico, uno spirito repubblicano, che noi dobbiamo ricreare dalle fondamenta e non per sua responsabilità, lei arriva alla fine di un percorso politico e istituzionale, lei non porta responsabilità esclusive su questo. Ma dalle grandi emergenze nazionali - e l'Italia del Novecento vi è passata perlomeno un paio di volte - si esce ricreando uno uno spirito di comunità larga, altrimenti è complicato superare crisi che abbiano caratteristiche che ci gettano dallo stato di emergenza a uno stato di eccezione e lo stato di eccezione ha bisogno di uno spirito repubblicano formidabile e lo spirito repubblicano si può ricreare, sì, grazie a una maggioranza parlamentare, ma - aggiungo io - perché non confidando in un tavolo istituzionale che coinvolga l'intero Emiciclo? L'hanno fatto prima di lei tutti coloro che sono passati da emergenze del genere.

perché è già successo più di una volta che comitato tecnico-scientifico da una parte e una parte del suo Governo siano entrati in rotta di collisione: penso e parlo di un problema che conosco abbastanza, quello dei trasporti. Il decreto ministeriale n. 39 del luglio scorso obbliga scuola e Ministero dei trasporti a mettersi in armonia, perché altrimenti non è possibile governare correttamente la riapertura delle scuole. E siamo di fronte ad un Ministro dei trasporti che non crede in ciò che vede, ma vede ciò che crede. Vedo che lei continua - ha fatto bene e condivido - finalmente a mettere il dito su questo punto, perché immagino, ascoltando il comitato tecnico-scientifico, che da lì siano germinati i punti di crisi più grande. Il rischio che vedo è che la coesione sociale e territoriale possa in qualche modo entrare in una crisi non dico irreversibile, ma che siamo obbligati ad affrontare con armi straordinarie. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, convocando poche ore fa il Consiglio supremo di difesa, il Consiglio supremo di difesa, un organismo istituzionale autorevolissimo, che si convoca in momenti particolari e lei lo sa bene. signor Presidente del Consiglio, colleghi senatori, è evidente che la forte diffusione dei contagi sta mettendo in ginocchio l'intera Europa e molti Governi del continente stanno assumendo provvedimenti duri e dolorosi. Se è chiaro, però, che la pandemia non è colpa dei Governi - e questo deve essere chiaro, se non a qualche bizzarra diciamo minoranza - e non è colpa neanche dei cittadini, dovrebbe essere altrettanto chiaro che i Governi, nel fronteggiare l'emergenza a mio avviso - dovrebbero dimostrare la stessa responsabilità e diligenza che pretendono dai cittadini. del Consiglio, da marzo dell'anno scorso l'attività legislativa del suo Governo non ha avuto tregua: un profluvio di decreti-legge,

Non ho l'impressione che il profluvio di questa attività legislativa sia pari all'efficacia. A mio avviso, siete arrivati alla seconda ondata, che qualcuno negava,

i trasporti e la scuola. Sono i settori dove, secondo me, l'impreparazione si è dimostrata più evidente. È saltato il tracciamento dei contagi, non sono state adeguate le strutture sanitarie territoriali e ospedaliere, a partire da quelle intensive, e abbiamo assistito a ore e ore di code di cittadini per fare un tampone.

speso giorni sui banchi a rotelle sì o banchi a rotelle, mentre, in realtà, mancano i professori e i presidi e le scuole non sono state sanitizzate. Ogni volta che si presenta l'occasione, lei e molti colleghi insistete e invocate il senso di responsabilità per il benessere del Paese, ricordando che siamo tutti nella stessa barca e avanti contando. E io, ogni volta, mi chiedo se questi appelli accorati si rivolgono anche alla sua maggioranza, in particolare al MoVimento 5 Stelle, o se loro, nel loro tetragono, irragionevole e puramente identitario rifiuto del MES, ne siano esentati per non troppe misteriose ragioni. infatti, quei soldi li avessimo presi il primo giugno, forse niente sarebbe al punto in cui si Quindi, è inutile rispondere con arroganza ai lavoratori dello spettacolo che protestano, perché non hanno piena consapevolezza della gravità della crisi - come ha detto un suo autorevole Ministro - perché non è così. Veramente non è così che si può chiamare tutti a quel senso di responsabilità che, a volte, non dimostrate neppure voi. Tralascio il rapporto con le Regioni: chi chiude, chi apre, chi chiude a metà e Io penso che il costo dell'impreparazione si aggiunge a quello della pandemia e lo rende più gravoso. Penso anche, presidente Conte, che ammettere di aver fatto errori o sottovalutazioni sia il modo migliore per meritare la fiducia per il nostro comune futuro. *(PD)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, rappresentanti del Governo, autorevoli colleghe e colleghi, siamo chiamati spesso a intervenire su temi complessi e difficili per il futuro del nostro Paese e per la salute dei nostri concittadini. Ogni volta ci deve tremare la voce, ogni volta dobbiamo essere preoccupati di usare termini e parole sbagliate. Ho deciso di essere come al solito franco, diretto, e parlare dal nostro punto di vista, quello del Partito Democratico, con grande trasparenza. Lo dico subito: il Partito Democratico, il Gruppo che ho l'onore di rappresentare, nel merito è a favore del decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri e concorda sui contenuti del decreto che avete varato nelle ultime ore, semplicemente perché il Paese aveva bisogno di questo. Avete dovuto farlo e noi apprezziamo che lo abbiate fatto nel modo migliore possibile.

i momenti di incontro, le occasioni di scambio del nostro peggior nemico, il virus. Lo avete fatto nei modi che avete ritenuto, seguendo le indicazioni

ovviamente vi invitiamo di nuovo a tornare in Parlamento a spiegarcelo, e noi saremo al vostro fianco con un obiettivo: esattamente come si fanno i DPCM

quando ci dice che il Governo e - aggiungo - il Parlamento devono fare di tutto affinché queste misure siano limitate nel tempo, e perché ciò avvenga è necessario che siano incisive.

ho espresso su questo un'opinione che confermo: tutto ciò mi sembra archeologia politica, guardandosi intorno, negli altri Paesi, in tutto il mondo, vedendo cosa sta succedendo. Credo che si debba essere coscienti del quadro che ci è dato vivere oggi e rispettosi della vita anche di ogni singolo cittadino che saremo in grado di salvare con questi provvedimenti. Ho sempre rispetto di chi esprime la propria libera opinione, anche nelle piazze, anche contro quello che sto dicendo io, ovviamente, o quello che sostiene il Governo. Ho, però, anche disprezzo - e sottolineo questo termine - per chi, in un momento come questo, spera di lucrare sulla più grande tragedia che sta vivendo il nostro Pianeta. Signor Presidente, non mi interessa al momento se sono stati fatti errori. Sono valutazioni che farà il corpo elettorale quando sarà chiamato a farlo, che faremo noi nelle discussioni parlamentari, nei Gruppi, che faranno le singole persone tra di loro.

mi interessa guardare al futuro del Paese. E, per guardare al futuro del Paese, ho delle richieste da farle: le chiedo, signor Presidente, Presidente, di valutare - lei, non altri, non gli opinionisti sui giornali - se i singoli Ministri siano adeguati all'emergenza che stiamo vivendo, questo è importante. Questo Governo deve andare avanti e deve avere le migliori donne e uomini che possano salvare il nostro Paese. Sempre a lei, signor Presidente, spetta la verifica - visto quello che si legge della tenuta della maggioranza. Noi dobbiamo contare su una maggioranza parlamentare solida che ci permetta di governare bene il nostro Paese. *(Applausi)*. Signor Presidente, è sempre a lei l'onere - forse l'onore, ma soprattutto l'onere in una fase così difficile di trovare il modo di coinvolgere le opposizioni. Ho chiesto di parlare tra i primi perché lo voglio dire alle forze di opposizione: certamente hanno posizioni diverse, di grande critica, non devono essere distruttive; devono valutare, quando fanno un intervento e dicono una cosa, se quell'intervento e quella presa di posizione fanno bene al futuro del nostro Paese e alla comunità nazionale. Ma devono avere un luogo, che sta a lei individuare, che sia una Commissione parlamentare bicamerale, che sia un'altra struttura, dove si possano confrontare con il Governo e con la maggioranza, che sia un comitato di salvezza nazionale. Permettetemi un inciso di richiamo ai nostri amici francesi. Comitato di salvezza nazionale mi ricorda «*liberté, égalité, fraternité*»: solidarietà da parte di tutto il Parlamento agli amici francesi e al presidente Macron per quello che è successo nelle ultime ore. Il coinvolgimento parlamentare, signor Presidente del Consiglio, è centrale. Il Parlamento rappresenta il Paese. I parlamentari tutti, di maggioranza e opposizione, hanno relazioni sul territorio. Il Parlamento va ascoltato, le istanze che provengono dal Parlamento sono un tesoro utile per l'azione di Governo. Ci avviciniamo alla legge di bilancio che, con i fondi aggiuntivi europei, sarà la chiave di volta di questa vicenda e di questa situazione. Non ci possiamo permettere di sbagliare, signor Presidente. Diamo la nostra disponibilità e chiediamo a tutti i colleghi e a tutte le forze politiche di collaborare. Se mostriamo di essere una comunità unita in questa fase e se saremo capaci, ognuno dalle proprie posizioni, di dare il nostro contributo, credo che usciremo da questa crisi, anche più forti e più capaci di dare speranza ai nostri cittadini. Questo è quello che oggi il Paese ci chiede: non polemiche, ma verità, responsabilità e futuro. Noi, signor Presidente, non possiamo sbagliare.

qualche tempo fa esistevano nell'Africa australe delle tribù che vivevano cacciando e utilizzando delle frecce imbevute di una sostanza velenosissima. A quelle tribù appartenevano tanti gruppi familiari diversi; eppure, ogni volta che bisognava decidere del destino di quel popolo, quelle tribù si sedevano a discutere. Per evitare che a qualcuno venisse in mente di usare quelle armi potentissime, avevano escogitato un metodo, in realtà molto pratico, che consisteva nel delegare un membro del gruppo a collezionare tutte le armi e nasconderle in un luogo sicuro fino a quando non fosse terminato il confronto. E così il gruppo si sedeva e discuteva anche per giorni, per notti, fino ad arrivare a una soluzione condivisa dei problemi. Oggi, il mio invito in quest'Aula è quello a deporre ciascuno le proprie frecce, le proprie differenze, e a lavorare tutti insieme *(Applausi)*, per portare questo Paese fuori dalla più grande crisi dal dopoguerra ad oggi. Sono momenti difficili per tutti. Da giorni ricevo messaggi di tutti i miei colleghi medici, che mi raccontano di nuovo di reparti sovraffollati, di carenza di posti letto, di turni massacranti. Allo stesso tempo, proprio qualche ora fa ho ricevuto il messaggio di un imprenditore, preoccupato di non riuscire a ripartire, perché la sua attività è stata nuovamente chiusa, nonostante avesse investito i risparmi di una vita per metterla in sicurezza. Sembrano posizioni inconciliabili, ma il nostro compito deve essere proprio quello di riuscire a trovare un percorso, che - come ha detto, signor Presidente - metta in sicurezza la salute e l'economia. Per fare questo, però, abbiamo un alleato preziosissimo, che ogni giorno muove passi da gigante, ovvero la scienza. Quando sono arrivata per la prima volta in quest'Aula, due anni e mezzo fa, dopo vent'anni trascorsi a occuparmi di scienza e di ricerca biomedica, prima a Washington e poi a Napoli, mi chiedevo spesso come parlare di scienza e di ricerca in quest'Aula e come sensibilizzare i miei colleghi sull'importanza di investire in questi settori. Mai avrei immaginato che avremmo parlato così tanto di scienza e di ricerca, perché, per la prima volta nella storia, stiamo prendendo decisioni politiche seguendo un metodo scientifico e questo - a mio avviso - è fondamentale. È solo grazie alla scienza se oggi riusciamo a intravedere una luce, al di là di questo buio.

che ci consentono oggi di fare diagnosi tempestive; abbiamo dei protocolli che riescono a rallentare l'evoluzione clinica della malattia; stiamo mettendo a punto farmaci antivirali e anticorpi monoclonali e quindi non bisogna perdere adesso la rotta. È fondamentale che le Regioni mettano in atto tutte le direttive ministeriali di riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete territoriale.

Per noi infatti è fondamentale programmare, avendo le idee chiare, e in questa programmazione dobbiamo mantenere vivo il ricordo di quello che abbiamo vissuto, il ricordo dei medici bardati negli scafandri, il ricordo delle bare di Bergamo. Manterrò vivo nel cuore il ricordo di Anna Maria, la mia collega di una vita, anche lei ricercatrice al CNR, che ad aprile mi ha lasciato per Covid *(Applausi)* e che ho provato per venti giorni a strappare al ventilatore che la teneva in vita. Mai come oggi, signor Presidente, questo ricordo è vivo, perché siamo ripiombati nello stesso incubo. Dobbiamo dunque pensare a una nuova normalità nuova normalità che, per, forza di cose, sarà fatta di didattica a distanza, di *smart working*, di ricette dematerializzate, di presa in carico territoriale e cura di prossimità. Forse serviva un virus per capire, a caro prezzo, che è possibile anche un'altra normalità. Noi però questa normalità, questo nuovo futuro dobbiamo essere bravi a saperlo costruire, partendo proprio dal mettere da parte le nostre differenze, le nostre frecce, e costruendo una rete di sicurezza che tuteli la salute e l'economia. È iscritta a parlare la senatrice Unterberger. Ne ha facoltà. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, siamo nella seconda ondata e, se qualcuno vuole dare la colpa al Governo, dovrebbe dare la colpa a tutti i Governi d'Europa: ha un milione e 200.000 contagi, i dati fuori controllo di Svizzera, Belgio e Olanda; la Francia costretta a un nuovo *lockdown*, per non dire poi di quello che succede nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Certo, mentre la prima ondata ci ha travolto come uno *tsunami*, la seconda era prevedibile e avrebbe dovuto essere preparata meglio. Ma anche questo però vale per tutti i Paesi europei e, soprattutto, non può essere contestato da chi, solo poche settimane fa, si rifiutava ostinatamente di portare la mascherina anche in Senato. Il virus si nutre di relazioni sociali e non ci sono ricette o verità assolute per debellarlo prima del vaccino. Tutti devono procedere per tentativi: lo fa la politica e lo fa anche la scienza, che non parla con una voce sola. Poi si può discutere se questa o quella misura era giusta o sbagliata, ma, tenendo ferma la volontà di non chiudere le scuole e le attività produttive, non rimangono molte scelte, anche perché non è vero che i trasporti pubblici possono essere facilmente potenziati, come oggi spiega bene il governatore Fedriga su «la Repubblica». Consiglio dei ministri sulla chiusura serale dei ristoranti e dei luoghi di svago sono un tentativo in atto un po' dappertutto, come primo passo per evitare misure più dolorose. Prendiamo per esempio la Germania, che ha uno sviluppo pandemico simile al nostro. Sappiamo che è uno Stato federale, dove la competenza per intraprendere le misure spetta solo ai *Land*. Ebbene, ieri la cancelliera Merkel, d'intesa con tutti i Presidenti dei *Land*, ha deliberato esattamente le stesse misure che sono contenute nel decreto del chiusura dei ristoranti e dei bar alle ore 18 e di cinema, teatri, palestre nonché di tutte le attività di svago alle quali si può rinunciare per prime. Stamattina si è tenuto il dibattito nel *Bundestag,* in cui la Merkel ha testualmente detto che sono misure necessarie, idonee e proporzionate. Pertanto, rimproverare al Governo italiano che le misure non si basano su dati scientifici mi sembra un po' tirato per i capelli. Naturalmente c'erano anche in Germania le critiche delle opposizioni e le stesse discussioni come da noi sul ruolo del Parlamento, sulla libertà individuale, sui trasporti e sulla mancanza di medici. Le critiche più ostinate sono arrivate dall'AfD, il partito che in Europa è alleato con la Lega.

siccome sappiamo che certe fasce della popolazione sono molto fragili e altre no, dobbiamo isolare solo quelle, perché - dice testualmente - la libertà vale di più della vita.

che così si ammazza l'economia; il giorno in cui si cerca di evitare una nuova chiusura, si obietta che così si gioca con la salute delle persone. scorso, quando ho criticato il Governo per l'approccio centralistico nella gestione della fase 2, dalle opposizioni ho ricevuto moltissimi applausi. Oggi che invece il Governo coinvolge di più gli enti locali, gli stessi dicono che si lava le mani e scarica la responsabilità su Regioni e sindaci.

Mi vanno bene tutti gli appelli a un maggiore coinvolgimento delle opposizioni, che credo sarà possibile però solo quando anche esse mostreranno un atteggiamento più costruttivo e responsabile. Se chiediamo ai cittadini di essere responsabili, dobbiamo esserlo per primi, altrimenti non stupiamoci che i più colpiti dalle misure protestino in piazza con la drammatica infiltrazione dei professionisti del caos e della protesta.

È bene coinvolgere maggiormente gli enti locali che, come abbiamo sempre detto in quest'Aula, sono quelli che hanno il polso della situazione, perché ci sono differenze da territorio a territorio.

Certo, la pandemia porta a galla la fragilità del sistema Italia, che vede una carenza strutturale di personale, medico, infermieristico e scolastico. caso, però, devo constatare che le critiche più feroci vengono proprio da quelle forze politiche che, con la loro misura di bandiera, quota 100, hanno aggravato questa situazione. La carenza di personale ospedaliero è sentita molto anche nel Sud Tirolo; molti dei nostri ragazzi che vanno a studiare nei Paesi di lingua tedesca restano poi lì per le migliori condizioni lavorative che vengono loro offerte. come abbiamo più volte contestato, i medici e gli infermieri che dalla Germania e dall'Austria vengono da noi, per via di un'assurda legislazione che contraddice lo spirito europeo, non possono lavorare nella nostra Provincia, nonostante la nostra popolazione sia per due terzi di madrelingua tedesca e per il 90 per cento perfettamente bilingue. Questo senza una ragione logica, se non per un nazionalismo fuori tempo, che un Governo di centrosinistra dovrebbe rifiutare.

serve davvero spirito collaborativo tra tutte le forze politiche e tutti gli attori istituzionali. Il nemico si chiama coronavirus, non dimentichiamocelo.

Alcuni ci dicono che non vorrebbero stare nei nostri panni di politici, perché dobbiamo assumere decisioni complicate e sofferte. Il suo discorso, signor Presidente, era intriso della sofferenza relativa alla difficoltà del momento.

«alle attività essenziali», ma all'umanità più profonda, a mettersi in relazione con l'altro, evitando abbracci, baci e incontri persino in famiglia, con figli e nostri amici, perché questa è l'arma per combattere il virus. È una prova durissima per la nostra profonda umanità. Di conseguenza andiamo a rinunciare alla nostra libertà personale, con il rischio, a causa di ulteriori provvedimenti restrittivi per proteggere la salute, di produrre nuovi disoccupati e di allargare ancora di più la forbice tra garantiti e non. Credo infatti, signor Presidente, che siamo tutti consapevoli che non esiste né in natura, né in un'altra ipotizzabile forma, alcun ristoro che compensi la dignità del lavoro, che costituisce l'essenza della soggettività umana e della persona. Non esiste alcun ristoro che compensi ed equivalga al fondamento della Repubblica democratica, il diritto che la stessa riconosce a tutti i cittadini. La drammaticità del quadro epidemiologico non è diversa né più grave della tragicità dello sconvolgimento sociale e psicologico nel quale la popolazione italiana versa e i fatti degli ultimi giorni ne sono testimonianza. Condanniamo gli episodi di violenza, ma mettiamoci in sintonia con il grandissimo disagio sociale della nostra popolazione. La tutela della salute deve essere allora in armonia con lo sviluppo dell'economia e del lavoro e dobbiamo assolutamente garantire il diritto alla scuola. La politica è fatica, perché è fatta di scelte di priorità. Due grandi Paesi, Francia e Germania, che si apprestano a decidere *lockdown* più o meno duri hanno una priorità: lasciare aperta la scuola. Perciò dobbiamo accompagnare e guidare quest'ora buia - per parafrasare il grande Churchill - con un piano concreto di qui a sei mesi, signor Presidente, o almeno a medio termine. È questo che chiediamo come Italia Viva. Quale luogo migliore per confrontarci tra parlamentari, di maggioranza e opposizione, e anche naturalmente tra partiti eterogenei, presenti nella stessa maggioranza? Dobbiamo mostrare la luce dopo il buio, perché nel 2021 dovremo riprendere a correre. Questa è la richiesta che le rivolgiamo: un confronto politico approfondito, serio, per non guardare solo al giorno dopo al prossimo DPCM, ma per traghettare la nostra Nazione oltre la crisi. La politica non è altro che una risposta ai bisogni della popolazione, quindi è nello stesso tempo celerità e lungimiranza. Allora, signor Presidente, non si arrabbi con noi; occorre che tutti tutti insieme facciamo in modo che l'apparato dello Stato e quello dei Ministeri non accumulino ritardi di alcun genere. Dobbiamo impegnarci giorno e notte affinché i vertici dell'INPS garantiscano che non ci siano mai più ritardi nell'erogazione della cassa integrazione e di altri sostegni affinché i Ministeri non accumulino altri ritardi. Faccio un esempio per tutti: abbiamo all'esame in Commissione un disegno di legge sui defibrillatori, approvato alla Camera, tanto atteso dalla popolazione italiana, che rimane fermo per le lungaggini dei pareri all'interno dei Ministeri. Questo, signor Presidente, in un momento di crisi non possiamo Per questo, priorità assolute sono per noi un sistema nazionale di tracciamento, di tamponi e di sorveglianza attiva, un progetto di prevenzione nazionale, la medicina territoriale e il MES.

Nessuno di noi può prendersi la responsabilità di non avere a disposizione altre risorse, tantomeno lei. Un appello finale, signor Presidente: tutto questo lo facciamo con una conduzione univoca e chiara del rapporto Stato-Regioni. Abbiamo 21 sanità diverse e in un tale assetto costituzionale abbiamo il dovere di avere una conduzione univoca tra Stato e Regioni, perché i nostri cittadini devono essere uguali e avere pari opportunità in tutto il territorio italiano. Il popolo italiano ha affrontato guerre, carestie e difficoltà sociali ed economiche, che ha superato sempre con uno spirito coeso e con la guida di classi dirigenti forti e coraggiose. Che anche questa volta la storia sia *magistra vitae*. Facciamo in modo, con

collega Castellone, l'abbiamo votato anche noi, mettendo via le frecce; ma quella riunione dura da nove mesi e credo che, a questo punto, le frecce si siano

il centro di ricerca dell'università di Oxford stima oggi che l'Italia è la peggiore d'Europa rispetto a quelli stanziati (non erogati). Presidente, a proposito di mettere da parte le frecce, è quello del «La mia esperienza finisce qui», con il governo Conte I: lo disse in quest'Aula, davanti a tutti noi. Lei è quello del bazooka da 400 miliardi, la potenza di fuoco. Lei è quello del ristoro dell'altra volta, il famoso fondo perduto, che ancora tutti stanno attendendo, perché non è arrivato;

che ristorerà un intero anno, ma poi si scopre che invece ristorerà il 100 per cento dell'ultimo ristoro, oppure fa riferimento, come per i locali di intrattenimento, agli incassi del mese di aprile. Chiunque sappia come funziona un locale di intrattenimento sa che nel mese di aprile i locali invernali hanno già chiuso e quelli estivi non hanno ancora riaperto. Lo sa anche un bambino.

dall'inizio dell'epidemia e purtroppo sono decedute migliaia di persone. Di fronte a questo, ognuno di noi interpreta il proprio ruolo

Vogliamo scommettere, signor Presidente, che a metà novembre non arriverà niente? La facciamo una scommessa io e lei, signor Presidente? Scommettiamo un caffè: uno per me, uno per lei e uno per

Oggi esistono questi due paradigmi, signor Presidente, che abbiamo ribattezzato, da un lato, contenimento e, dall'altro, mitigazione. Dobbiamo riscrivere il dizionario dei sinonimi e dei contrari. per farci capire da chi ci ascolta, è la parte che dovrebbe fare lo Stato (quello con la S maiuscola), mentre la mitigazione è la soppressione è la soppressione delle libertà d'impresa e di movimento, la coercizione delle attività commerciali

condizioni estreme, quali erano quelle di marzo e di aprile, non oggi, che sono passati nove mesi, durante i quali abbiamo fallito ogni operazione sull'altro versante, quello del contenimento.

in diretta a ogni DPCM, non si fidano di lei e non credono alle sue misure. È per questo che non scaricano l'*app* Immuni; hai voglia a fare pubblicità progresso, con Fedez e *company*.

il professor Brusaferro. Oggi stiamo di nuovo ragionando sulla necessità di tracciare gli asintomatici, perché questo è lo scrimo, la linea del Piave: riuscire a scoprire chi non ha sintomi e

non più tardi di ieri. Oggi lei ci dice che finalmente, dopo che il sottoscritto (insieme a tanta altra gente, evidentemente) ha ribadito per mesi la necessità di fare centinaia di migliaia di test,

Tutte queste cose andavano fatte prima, non adesso, e l'avevamo detto. Collega Unterberger, si è intrattenuta dicendo che non ci sono proposte da parte dell'opposizione, ma non può non ricordare quante volte abbiamo parlato in quest'Aula; ha votato insieme a me una mozione unitaria che prevedeva di fare tamponi a tappeto. O forse non l'ha letta e non se n'è accorta?

c'è un'inappropriatezza diffusa, sia nell'ospedalizzazione, in entrata e in uscita, sia nelle cure domiciliari. Non c'è un protocollo a beneficio dei sanitari, dei medici di medicina generale e degli ospedalieri, che detti

alla percezione di insicurezza sanitaria che purtroppo prende alla gola i nostri concittadini - ne sono riprova gli atteggiamenti che tutti censuriamo, ma comprendiamo

In combinazione con la percezione di insicurezza sanitaria, quella di ingiustizia, che in questo momento trapela, può determinare danni gravi alla nostra convivenza civile. e ci dice che questo è il momento di restare veramente uniti. Bene, allora la faccia un'operazione per restare veramente uniti:

È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

troviamo pertanto di fronte, ancora una volta, a una situazione molto complicata e difficile. Il Governo ha assunto, di volta in volta,

tutti - a questo punto della situazione serve ancor di più una programmazione strategica,

Questo sport dello scaricabarile è francamente intollerabile. Abbiamo assistito addirittura, ieri, ad un Presidente di Regione che si è messo a manifestare insieme

abbiamo ripetuto varie volte - e ora bisogna farlo - di rafforzare i servizi medici territoriali e anche i medici di base. Infatti, non è che il Governo non volesse fare le convenzioni con i medici di base; ci sono state, anche in quel caso, chiusure molto forti.

alle questioni che stanno appassionando tutti, come i piani regolatori degli orari delle città. Lo devono fare obbligatoriamente

traguardano il contenimento del virus, sapendo tutti che questa pandemia avrà un finale che nessuno di noi conosce e che soprattutto sarà quello vero quando ci sarà il vaccino e quando lo potranno utilizzare tutti. Quindi nessuno è in grado, oggi, di programmare questo finale.

un'assenza di programmazione e di capacità di decidere che le priorità che mettiamo al centro sono intrecciate con l'insieme delle condizioni di vita e di lavoro, di costruire davvero da subito le condizioni di intreccio di interventi e di investimenti, avendo anche la possibilità di finanziamenti europei,

mio parere altrettanto bella: «Il mondo è un posto pericoloso non per quelli che compiono azioni malvagie, ma per quelli che osservano senza fare cose e per quelli che fanno cose senza saperle fare». Noi glielo abbiamo detto fin dall'inizio: di fronte a una pandemia, di fronte a un mostro mellifluo che sta mettendo il mondo in ginocchio da marzo, si faccia aiutare. Non si faccia travolgere dalla tentazione dell'uomo solo al comando. Non creda, a livello comunicativo, di poter governare un'opinione pubblica per sempre. Non è possibile, al netto dei contenuti. Non perché glielo diciamo noi: glielo sta dicendo la sua maggioranza. Ha appena detto cose importanti. Noi abbiamo ascoltato e condividiamo da sempre il fatto di poter collaborare, ma non per avere seggiolini, strapuntini, posticini in Commissione o Presidenze di Commissione. Non è quello che ci interessa, presidente Conte. *(Applausi)*. Noi, a partire da marzo, le abbiamo proposto delle ricette, le abbiamo dato delle soluzioni, le abbiamo detto quali erano le pietre d'inciampo di questa pandemia: e sono ancora quelle. Lei ha detto che mantenere lo stato di emergenza ha aiutato il Governo a governare e a gestire la crisi. Non è vero. Se così fosse, se lo stato di emergenza avesse funzionato e le cose fossero andate bene, a cosa si dovrebbero imputare quei dieci chilometri di code che abbiamo visto davanti ai Pronto soccorso, con una medicina d'urgenza

sbagliato sulla *app*, un mancato investimento sui tracciatori, che non sono mai esistiti. Ebbene, se qualcuno sciaguratamente incappa in un tracciamento della *app* Immuni, è costretto a rimanere chiuso in casa in libertà vigilata a tempo indeterminato perché non riesce a fare un tampone privatamente. Questo è il modo in cui lei ritiene lo stato di emergenza abbia funzionato? Lei ci ha detto a luglio che aveva bisogno di leggi speciali per governare l'Italia, ma neanche quelle sono servite. Signor Presidente, non è riuscito a governare la situazione. Per quale motivo? E la prego di non fare gestacci, non è urbano da parte sua fare gestacci in Parlamento;

è veramente la pietra di inciampo, non di questo Governo ma degli italiani, di tutti quelli che stanno affrontando una seconda ondata che eravamo perfettamente consapevoli sarebbe arrivata. Lo sapevate anche voi. Noi ve lo stiamo dicendo da aprile. Vi abbiamo proposto di aprire ospedali Covid ogni 500.000 abitanti; vi abbiamo dato dei suggerimenti molto concreti; vi abbiamo dato dei documenti, che non so dove lei abbia messo e non so se li abbia mai letti. Vi avevamo detto che sarebbe stato pericoloso combinare l'emergenza Covid con l'emergenza influenzale ordinaria. Dove sono i vaccini antinfluenzali? Le sembra compatibile con uno stato di emergenza che ha funzionato quella coda di persone anziane che noi vediamo alla ricerca disperata di vaccini antinfluenzali che non ci sono? Io le sto parlando molto pacatamente. Sono molto più pacata della sua maggioranza, che le ha lanciato dei segnali molto forti. Anzi, se mi posso permettere, anziché lanciarvi messaggi in Aula, scrivervi lunghe lettere sui giornali, telefonatevi; telefonateci. Noi ci siamo e siamo sempre disponibili alla collaborazione. L'importante è che ci ascoltiate. *(Applausi)*. Abbiamo parlato di scuola. Colleghi, voi mi siete testimoni: quante volte, tutti noi di Forza Italia, della Lega e di Fratelli d'Italia vi abbiamo parlato di scuola vi abbiamo pregato di affrontare il tema scuola in maniera professionale? Non dico altro. Troppe cose abbiamo detto e tante altre cose vi diremo. Un'unica immagine: in questi giorni voi state consegnando i famigerati, famosi, costosissimi banchi a rotelle nelle scuole chiuse! Non c'era modo di impiegare diversamente questi soldi, magari per rimpolpare quelle piante organiche di medici, e infermieri che adesso state chiamando? Non a giugno, a luglio, ad agosto o a settembre: adesso li state chiamando. Adesso state facendo i concorsi per le terapie intensive. Questo lei lo chiama stato di emergenza? Mi perdoni, glielo dico molto laicamente, ma io non sono d'accordo su questa gestione. Ve lo abbiamo detto in ogni modo possibile e lei non lo sa oggi dalle mie parole: lei lo sa da tutte le cose che abbiamo continuato a dirle in questi sette mesi in questi sette mesi e tutti noi, come opposizione responsabile, abbiamo il dovere di ricordarglielo. Ripeto, lei, come Governo, ha il dovere di renderci conto di questi ritardi. Perché non sono state fatte queste cose? Perché? Cosa si aspettava a fare le terapie intensive? Si sapeva che ci sarebbe stata la seconda ondata e ora anche la terza, ma non mi voglio ripetere. Lei sicuramente sente il rumore della piazza, e non della piazza cattiva, quella dei contestatori professionali, dei disturbatori; no, la piazza della gente che ha paura di chiudere per non riaprire mai più! La piazza degli esercizi commerciali, quelli che hanno fatto tutto in regola, che hanno speso soldi fino a

È ovvio che si sentano traditi, è ovvio che siano in piazza: hanno ragione, anche perché il problema è stato affrontato dalla coda. Signor Presidente, lei lo sa, ci ha gentilmente consultato dieci minuti prima di emanare il DPCM, però, glielo dico con affetto, se per caso ci chiamerà cinque minuti prima per dire che chiude l'Italia noi le attaccheremo il telefono. Questa volta basta! Signor Presidente, il DPCM prende il problema dalla coda. Perché non avete deflazionato il trasporto pubblico locale? Gliel'ha detto un suo coordinatore del comitato tecnico-scientifico, quello che lei invoca ed evoca sempre, il professor Miozzo, il quale ha dichiarato che è da aprile che dice al Presidente del Consiglio che deve fare una stretta sui trasporti. Ed è evidente che quello su cui si deve agire non è il commerciante virtuoso che si è messo in regola, ma il mezzo di trasporto dove ci si contagia perché ci sono "sardine" strette tra di loro - anche se mascherate - che si trasmettono il virus. *(Applausi).* E questo vale per gli autobus, le metropolitane, le corriere, gli aerei

Signor Presidente, la prego, non è troppo tardi, però non facciamo più demagogia sulla pelle degli italiani, quelli che la stanno chiamando dalla piazza, quei contestatori che il Ministro dell'interno ha chiamato «autonomi». Vorrei fosse chiaro che sono «autonomi» da intendere come partite IVA, non come autonomi contestatori, partite IVA, non garantiti, perché il Covid non è una livella: ha diviso il mondo tra garantiti, che prendono comunque lo stipendio, la pensione o la cassa integrazione, e partite IVA, autonomi, professionisti, commercianti, che non prendono niente.

ci sono anni e anni di sacrifici, di spese, di bollette, di mutui, di burocrazia inutile, di tasse comunali, provinciali, regionali, statali, con delle sigle impronunciabili e urticanti. Oltre a tutto questo, adesso devono chiudere. Non le chiediamo provvedimenti folli, non le chiediamo l'incoscienza; le chiediamo la coerenza. Le chiediamo prima di tutto di collaborare, ma farlo veramente; lo ha detto il Capogruppo del Partito Democratico. Per noi - ripeto -collaborare vuol dire fare le cose insieme, non avere regalini o strapuntini; vuol dire condividere il contenuto dei provvedimenti, significa fare come, secondo noi, le cose vanno fatte per fare in modo che il nostro Paese affronti questa pandemia con armi migliori e non con le armi spuntate che in questo momento sono state proposte.

Va bene, però, signor Presidente, la prego: gli *stop* *and go* stanno ammazzando il Paese. Lo ha detto il presidente Berlusconi tempo fa: non possiamo sopravvivere al Covid e poi morire di fame. Tutti noi dell'opposizione lo impediremo in ogni modo possibile.

Signor Presidente, innanzitutto ritengo doveroso - so che il Senato l'ha già fatto stamattina, penso

Stiamo combattendo una malattia virale, ma intanto altri tipi di contagi non si fermano. Quindi siamo tutti francesi, senza se e senza ma da questo punto di vista. Signor Presidente Consiglio, è preoccupante che, in un momento così grave per il Paese, non ci sia uno scontro opposizione-maggioranza: state facendo tutto voi. Mentre in Italia cresce lo scontro sociale, abbiamo sentito in quest'Aula la bocciatura nei suoi confronti non dalle opposizioni ma dalla sua maggioranza *(Applausi)*, che in un momento così delicato arriva a chiedere un rimpasto di Governo. un rimpasto di Governo. Traduco dal linguaggio del PD e del collega Marcucci, che le chiede - e questo è allarmante - se tutti i suoi Ministri siano all'altezza della situazione. Evidentemente, se c'è una domanda, c'è anche una risposta: è evidente che un ministro come la signora Azzolina non è in grado di gestire la scuola italiana. *(Applausi)*, non è in grado di dare risposte agli studenti e agli insegnanti. Però risolveteveli nelle riunioni di maggioranza i vostri problemi interni. Le dico anche che il centrodestra è pronto a collaborare, ma non vogliamo e non ci interessa mezza poltrona. Vogliamo dare idee. Commissioni bicamerali no, non ci interessano. Il Paese ha già dato un responso chiaro, quindi la sfiducia nei suoi confronti non è del Senato, ma ma del Paese. Non abbiamo mai sentito una parola magica, che costa poco però dà la dimensione di una persona, in questi mesi e neanche oggi: «scusa». Non abbiamo sentito qualcuno dire: «scusa». Cosa avete fatto per sei mesi? i lavori negli ospedali, grazie a quel genio del commissario Arcuri, che lei, dopo i disastri per le mascherine e per la scuola ha nominato a sovrintendere la salute degli italiani,

domanda è: che cosa avete fatto a maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, oltre che ad occuparvi di banchi con le rotelle e monopattini? *(Applausi)*. Perché non vi siete occupati e preoccupati di ospedali? Sono fermi da giugno 400 milioni di euro per comprare nuovi autobus da Roma a Milano, da Torino a Napoli, perché manca una firma in un Ministero. Sono fermi nelle casse del Governo 80 miliardi di euro. Lei oggi viene ad annunciare il decreto ristoro per novembre-dicembre, le posso chiedere sottovoce di pagare i decreti di luglio, agosto, e settembre, che sono ancora fermi perché siete incapaci di passare dalle parole ai fatti? *(Applausi)*. Prima di promettere altri soldi, pagate quelli che dovevate. La cosa surreale è poi che un cittadino a casa pensa che il Parlamento si stia occupando da settimane e da mesi, giorno e notte dal lunedì al venerdì, di questa emergenza sanitaria, sociale, culturale ed economica. ieri la Camera si è occupata di omotransfobia; il dibattito giornalistico è occupato dalla legge elettorale. Avete passato un'estate a smontare i decreti sicurezza

Le proposte le abbiamo sentite, da parte degli amici di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, ma non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, magari perché parla un'altra lingua in quest'Aula. Quanto alle

non è un ennesimo *lockdown*, la chiusura totale, che sarebbe la sconfitta non tanto di Conte, di cui ci interessa poco, quanto dell'Italia e dell'economia italiana. Dobbiamo fare di tutto per evitare un'altra chiusura, e facendo cosa? Andando a curare le persone a casa loro usando tutti i mezzi e tutte le terapie necessarie, anche quelle che non piacciono alle multinazionali del farmaco perché costano troppo poco. lei ci ha annunciato come se fosse un gran risultato che i tamponi a domicilio sono frutto di un accordo che avete fatto questa settimana. Questa settimana? A fine ottobre? Ma voi sapete che, grazie al fatto che avete perso sei mesi di tempo, i lavori nelle terapie intensive non si faranno, perché,

Arcuri si dovrebbe dimettere oggi! In qualunque Paese normale, un commissario che fallisce si dimette, non viene promosso! Ma lei, più incapaci sono e più li promuove? È bizzarra questa cosa qua!

Se sugli autobus e sulle metropolitane non siete intervenuti, prendetevi le vostre responsabilità! Non contestiamo la chiusura di alcune attività economiche, se serve a salvare vite, ma mi spieghi che vite si salvano, chiudendo palestre, piscine, cinema e teatri che erano fra i più controllati e sicuri al mondo. *(Applausi)*. Che vite si salvano? Semplicità! Altra proposta: avete rinnovato per alcune settimane la cassa integrazione. Signor Presidente, glielo chiedono i consulenti del lavoro, i fiscalisti, gli avvocati e i commercialisti. Oggi, grazie alle vostre scelte bizzarre, ci sono 25 modalità operative diverse per accedere alla cassa integrazione. Semplificate la vita agli italiani, altrimenti fate decreti di notte che poi finiscono nel nulla di giorno. Lo dico a chi ci sta seguendo da casa, con enorme pazienza: delle chiacchiere degli ultimi nove mesi, il 90 per cento è rimasto aria fritta, perché si stanno aspettando 110 decreti attuativi per le promesse che avete fatto agli italiani. Non basta il titolo! Poi uno si stupisce se protestano a Napoli, a Verona, a Roma, a Milano, a Palermo o a Bergamo. Sono persone perbene: gli imbecilli, quelli con il volto coperto, con il casco e con il bastone in mano stiano a casa, perché la violenza non è mai la risposta e non è mai la soluzione sempre che non venga alimentata da qualcuno a cui conviene che nelle piazze ci siano dei violenti. Quindi non stupiamoci del fatto che la gente chieda risposte. Ci sono decine di scadenze fiscali non prorogate per novembre. Signor Presidente del Consiglio, almeno queste possiamo bloccarle e non rinviarle? Questo è un Governo fondato sui rinvii! Rinviamo le decisioni su Alitalia e su Autostrade ricordo che gli unici che hanno guadagnato dal caos autostrade sono i signori Benetton, alla faccia di quelli che chiedevano certezza della pena e del diritto! Ieri, signor Presidente del Consiglio - non sei mesi fa - la sua litigiosa maggioranza - Renzi ce l'ha con lei, il PD ce l'ha con Renzi, la Bonino ce l'ha con il mondo, in un tutti contro tutti che non ci possiamo permettere in questo momento -che la sostiene - vedremo per quanto tempo - ha bocciato un emendamento delle opposizioni che chiedeva una cosa normale, ovvero che lo Stato paghi i suoi debiti nei confronti delle famiglie e delle imprese italiane. *(Applausi)*. Sono 50 miliardi Quindi, prima di fare la morale agli altri, guardiamo in casa nostra. Passo all'ultima riflessione. Errare è umano perseverare diabolico, Presidente. A febbraio e marzo scorsi l'improvvisazione poteva essere accettata perché era una prima volta. Sono passati sette mesi non venite adesso a dirci che, nel nome del virus, chiudete teatri e ristoranti e fate uscire dal carcere 5.000 delinquenti che tornano a casa loro. *(Applausi)*. L'abbiamo già provato e non funziona. Gli italiani chiusi in casa e i delinquenti tranquilli a guardare le sue dirette su Rai 1! Quindi, noi ci siamo, non per i posti, che non ci interessano. Lei e i suoi parlamentari chiedete collaborazione,

Non è più il momento di specchiarsi e dirci quanto è bravo e bello. Sul canone estetico non intervengo, mentre sulla bravura una nuova chiusura significherebbe il fallimento di questi sei mesi di nulla da parte sua e del Governo. Noi siamo disposti a lavorare per salvare vite e posti di lavoro. Spero che nessuno sia disposto a lavorare per salvare se stesso e la sua poltrona, perché questa è l'impressione che ci date. Buon lavoro.

Potremmo quindi ricordare solo alcune piccole cose. Siccome si è sentito molto parlare di trasporti e sanità, ricordiamo di chi sono le competenze in questi ambiti. Mi sembra che siano delle Regioni, se non ricordo male. E mi sembra, oltretutto, che molte di queste Regioni siano governate dal centrodestra. Quindi, prima di parlare di quello che viene addebitato al Governo, è meglio guardarsi in casa propria e assumersi le proprie responsabilità.

quando aumenta la temperatura. Quindi, una prima cosa che dobbiamo fare per diminuire il livello di caos è raffreddare il sistema. *(Applausi)*. Questo significa agire e ragionare con lucidità e freddezza, perché la politica deve assumersi la responsabilità utilizzando il raziocinio, che non è naturalmente disgiunto dal cuore. L'entropia l'abbiamo vista anche in quest'Aula, in cui mi sembra che ci sia

E qui dobbiamo stare molto attenti a quello che facciamo perché quando ci troviamo di fronte alla necessità di compenetrare la salute delle persone con la loro libertà dobbiamo ricordarci di una cosa. Ancora una volta mi tocca citare il presidente Pertini, quando diceva che non c'è libertà senza giustizia sociale. Siccome ci troviamo nella condizione che per salvaguardare la salute delle persone abbiamo dovuto fare una restrizione del livello di libertà, dobbiamo parimenti aumentare il livello di giustizia sociale e in fin dei conti è quello che è stato fatto decreto-legge pubblicato oggi, in cui si affronta il tema e si cerca di riportare un livello di giustizia sociale accettabile per la vita delle persone. Ovviamente questo non ha fatto altro che accentuare un sistema che già c'era. Come tutti sappiamo, il sistema neoliberista ha esasperato le disuguaglianze. Abbiamo visto cosa è successo nei Paesi di lingua anglosassone, Stati Uniti per primi. Quindi ci troviamo in una condizione che è preesistente, con un aumento delle disuguaglianze e noi dobbiamo intervenire proprio per combattere questo enorme livello di disuguaglianza e fare in modo che ci sia un riequilibrio tra chi tanto ha e chi poco ha. Quindi dobbiamo ancora una volta pensare che dobbiamo far pagare le tasse a chi tanto ha, anche se magari sono società estere o anche se sono società che hanno acquisito molta più ricchezza in questo periodo, e cercare quindi di riequilibrare per dare al popolo quello di cui ha bisogno. La senatrice Bernini diceva che non bisogna morire di fame; chi può essere in disaccordo? Però, per non morire di fame, dobbiamo capire di cosa stiamo parlando.

credito d'imposta sugli affitti, cancellazione della seconda rata IMU, misure per i lavoratori dello spettacolo e del turismo, fondi di sostegno per alcuni settori più colpiti, proroga del reddito di emergenza e così via. Ci troviamo però anche nelle condizioni di vedere cosa succede in Francia e in Germania. In Francia il presidente Macron ha annunciato che da domani passeranno al *lockdown*; una cosa però non la faranno: non chiuderanno le scuole. Come ci ha detto il presidente Conte, l'istruzione è un valore irrinunciabile quindi noi dobbiamo mettere al centro il valore dell'istruzione, capire che non possiamo agire nella chiusura delle scuole e quindi intervenire nei confronti di alcuni pezzi

si è trovato a gestire una situazione incredibile, per posizionamenti che non vanno da nessuna parte. *(Applausi).* Il senatore Salvini ha detto che non vuole avere mezza poltrona; forse ne vuole avere una intera.

una nuova finestra"). L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, noi sappiamo che lei non è una fata e non può avere la bacchetta magica per risolvere con un solo tocco tutti i problemi dell'agricoltura che sono ovviamente antecedenti alla crisi del Covid. Possiamo dire, però, che è stata un po' timida nell'affrontare le tante questioni aperte. Per quanto riguarda il nutri-score, ad esempio, se non fosse stato il Gruppo Fratelli d'Italia a sollevare in Aula il problema, dopo averlo fatto con le etichette a semaforo o con la questione relativa ai pesticidi, il tentativo dei Paesi del Nord e delle grandi multinazionali di discriminare i nostri prodotti nazionali come il grano e il prosciutto sarebbe passato quasi sotto traccia. Quello a cui stiamo assistendo, infatti, signor Ministro, è un vero e proprio attacco alle nostre produzioni, la cui riconosciuta

Possiamo dirle che non ha certo affrontato e risolto il problema dei prezzi dei prodotti agricoli che troviamo sugli scaffali della grande distribuzione a prezzi addirittura inferiori ai costi di produzione. È ora che si lavori, Ministro, per un prezzo minimo garantito che dia dignità non solo ai braccianti, ma anche agli imprenditori. Ministro, le ricordo la concorrenza sleale, l'*italian sounding*, gli accordi commerciali europei che non tutelano il prodotto italiano mentre noi chiediamo da tempo l'introduzione dei dazi di civiltà nei confronti di quelle merci che provengono da quei Paesi in cui non si rispettano gli standard salariali, di sicurezza sul lavoro di tutela ambientale. È proprio l'agricoltura italiana che paga il prezzo più alto di questi accordi. È in questo contesto, già fragile e complicato, che il Governo di cui lei fa parte ha risposto con la chiusura di tante attività che sono uno sbocco naturale per molti operatori agricoli. Infatti, Ministro, i locali che il Governo ha chiuso costituiscono solo la punta dell'*iceberg* dell'intera filiera, che era stata messa già pesantemente in difficoltà nella prima andata, in cui lei e il suo Governo avete dato risposte più ideologiche che concrete, più di facciata che sostanziali. Le chiediamo pertanto se abbia contezza che questa crisi la pagherà l'intera filiera, con stime che le associazioni di categoria hanno già provveduto a fare, ma anche se non ritenga inutile e privo di evidenze scientifiche un DPCM che dà il colpo di grazia a tante realtà economiche che costituiscono oggi gli ambasciatori del *made in Italy*, l'eccellenza italiana nel mondo.

come Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, mi sono impegnata fin al giorno del mio insediamento per difendere, sostenere e promuovere, a livello nazionale ed europeo, il patrimonio agroalimentare italiano in tutte le sue declinazioni. È stato e continua ad essere il mio obiettivo principale. Ritengo non possa essere messa in discussione la mia attenzione e consapevolezza sul riacutizzarsi dell'emergenza sanitaria e sulle gravi ripercussioni a danno del sistema produttivo e occupazionale. È tra le ragioni per cui prosegue ininterrotto, anche in questi giorni, il confronto con le associazioni di settore e l'intera filiera istituzionale per avere dati costantemente aggiornati sulle ripercussioni del diffondersi del Covid-19 sul nostro comparto. Non è un caso che tra quelle indicate dagli interroganti compaiano le rilevazioni Ismea. Tale consapevolezza mi ha spinto a lavorare con la forza necessaria per ottenere gli stanziamenti utili ad attenuare e se possibile anticipare le conseguenze di una crisi che, se non adeguatamente governata, rischia di provocare fratture economiche e sociali difficilmente ricomponibili. La dialettica all'interno del Governo è nota; così la mia posizione, rivolta a trovare equilibrio e bilanciamento tra le esigenze di carattere sanitario e quelle di natura economica. Ma qui oggi conta restituire il lavoro in atto e le misure di merito rivolte alla filiera agroalimentare. Sotto questo ultimo profilo, giova ricordare che quest'anno, per i settori agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, abbiamo stanziato risorse pari a circa quattro miliardi di euro. Cifre prima inimmaginabili, ma che oggi si rivelano indispensabili a garantire liquidità e sostegno alle imprese che, con grande sacrificio, si stanno adeguando alle stringenti misure di contenimento. Tra le numerose misure adottate, voglio segnalare il decreto attuativo del *bonus* ristorazione, con cui destiniamo 600 milioni di euro di aiuti immediati alle attività di ristorazione che hanno acquistato prodotti agricoli e agroalimentari italiani. Una disposizione importante per il canale ho.re.ca, che io considero settore strategico della nostra economia e parte integrante della filiera agroalimentare. Vengo all'ultimo punto. Nel decreto-legge ristori, pubblicato oggi in *Gazzetta Ufficiale*, assicuriamo per il mese di novembre l'esonero contributivo, previdenziale e assistenziale per i datori di lavoro delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni. A questa misura, che vale oltre 350 milioni di euro, si affianca la costituzione di un fondo da 100 milioni di euro per sostenere, con contributi a fondo perduto, quelle imprese agroalimentari maggiormente coinvolte dalle limitazioni dell'ho.re.ca. Non nascondo come il lavoro da fare sia molto difficile e complesso, a maggior ragione perché sono assolutamente convinta che tutela della salute e salvaguardia dell'occupazione e del reddito delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese debbano andare di pari passo. Anche per questo considero importante l'apporto di quanti, tra le opposizioni, vorranno contribuire a migliorare i provvedimenti in un confronto leale, fattivo e virtuoso.

sia assolutamente fuori luogo. È infatti questo il luogo nel quale vengono messe in discussione proprio le politiche che un Ministro attua; questo è il tema e il fulcro della democrazia. Vorrei rileggerle quanto lei stessa dichiarò ai giornali, al quotidiano «La Stampa»: «Sabato ho ribadito per tutta la giornata come la chiusura dei ristoranti alle 18 fosse sbagliata». Continua dicendo: «Lo stesso comitato tecnico-scientifico avrebbe avanzato dubbi sull'utilità della chiusura. Chi ha fatto sforzi per mettersi in regola non deve sentirsi tradito». Ma la realtà, signor Ministro, è ormai che questo giochino del poliziotto buono (lei) e del poliziotto cattivo (Conte) lo hanno capito tutti; abbiamo capito quanto strumentale sia per cercare di mantenere la visione del Governo e la visione di una minoranza interna nello stesso perimetro, quello della sua maggioranza. Ministro, non funziona più. Lei è organica a questo Governo adesso, così come lo era quando, usando l'agricoltura, perorò ed ottenne la sanatoria per i migranti. Una sanatoria in linea sicuramente con il suo pensiero e con il suo percorso, ma non certo utile, come si è dimostrato, alla risoluzione dei problemi dell'agricoltura, che chiedeva tutta *voucher* e corridoi verdi. Oggi la proposta del Governo, venduta come la panacea di tutti i mali, sono i ristori. Ristori per rimediare a un vostro errore, quello delle chiusure senza evidenza scientifica che ne dimostri l'utilità. Tale errore ha precisi responsabili: voi, appunto. Indebitate ultimamente gli italiani oggi per rimediare a un vostro errore; lo Stato costringe a chiudere chi per legge si è impegnato ad adeguare i locali e a rispettare le leggi e i protocolli. Ma uno Stato che per decreto riduce o azzera le entrate di un'impresa, per essere serio e concreto deve intervenire sui costi fissi: sugli affitti, sui dipendenti, sui mutui, sulle utenze e sulle tasse. Non ci sono bonus e ristori che tengano, anche perché parlavate di un rimborso pari al 100, 150 o 200 per cento del calo del fatturato. Invece ci siamo svegliati tutti con un bonus del 100, 150 o 200 per cento del bonus previsto dal decreto rilancio. Costringete migliaia di imprese a chiudere per decreto. E allora, signor Ministro, a poco conteranno le sue parole di distinguo. E se le sue parole «siamo a pieno titolo nel Governo e ci resteremo fino a quando avrà senso per la qualità delle politiche che vengono messe in campo» hanno un valore, signor Ministro, delle due l'una: o lei ha usato questa frase per prendere in giro ancora una volta gli agricoltori e gli italiani oppure lei è ancora in questo Governo perché ne condivide la linea.

premessa che il repentino innalzamento della curva dei contagi da Covid-19, che ha portato all'emanazione degli ultimi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, non può esimere da una riflessione maggiormente approfondita sulle condizioni sanitarie ed economiche in cui attualmente versa tutto il settore dei trasporti, in particolar modo il settore del trasporto pubblico locale, e sulle garanzie di sicurezza per gli utenti. Dopo la ripresa delle attività scolastiche, si sono verificati folti assembramenti, soprattutto nelle grandi città, e non solo nelle ore di punta. Alle fermate della metropolitana

risultano ancora molto preoccupanti. Noi di Italia Viva-PSI riteniamo essenziale, per un'efficace azione di contrasto all'esponenziale aumento dei contagi, Presidente del Consiglio dei ministri, ma uno specifico piano di riorganizzazione dell'intera rete dei trasporti su tutto il territorio nazionale, che tenga conto delle differenze che attengono alle varie modalità di trasporto e ai mezzi. Considerato che lei, nei tavoli convocati al Ministero, ha confermato la decisione di mantenere il livello massimo dell'80 per cento di capienza raggiungibile all'interno dei mezzi di trasporto, che alcune Regioni come la Toscana hanno attuato misure più stringenti rispetto a quelle messe in atto dal Governo, oltre ad aver aumentato i servizi di trasporto aggiuntivi e alla luce del peggioramento della situazione epidemiologica, è evidente che queste misure sono essenzialmente da rivedere e da potenziare, ma soprattutto da condividere. Tutto quanto premesso, chiediamo di sapere quali siano gli orientamenti prossimi del suo Ministero rispetto alle problematiche descritte in premessa premessa e, qualora ne abbia conoscenza, le motivazioni che hanno determinato l'aggravarsi della situazione di criticità in cui versa il sistema trasportistico. Chiediamo altresì di sapere quali siano le ulteriori misure previste e le scelte che vorrà attuare, mi auguro in condivisione non solo con il Parlamento e con le Commissioni competenti, ma anche con gli enti territoriali e le rappresentanze del settore, per superare questa situazione incerta, che coinvolge i mezzi e le reti del trasporto pubblico e che rischia non solo di ledere il diritto dei cittadini di usufruire di servizi di trasporto una buona qualità, ma anche di causare forti preoccupazioni riguardo la corretta tutela della salute dei cittadini stessi e la tenuta del sistema Paese nel suo complesso.

tali da evitare il sovraffollamento dei mezzi nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza degli utenti, sono in capo alle Regioni in forza del Titolo V della Costituzione, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 32 della legge n. 833 del 1978.

vigenti, definite sulla base dell'analisi dei flussi puntuali della domanda di trasporto elaborata dall'Inail e oggetto di specifica condivisione con il comitato tecnico-scientifico, come da richiesta delle stesse Regioni, e con i titolari dei servizi di trasporto pubblico locale e responsabili dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico dedicato. Un percorso di condivisione, con Regioni ed enti locali. Nel corso della riunione di monitoraggio, le Regioni, le Province e i Comuni hanno evidenziato di aver provveduto ad incrementare i mezzi per le tratte con maggiore domanda, utilizzando 120 dei 300 milioni di euro messi a disposizione dal Governo con il decreto n. 111 del 2020, che hanno consentito l'utilizzo di 2000 mezzi di trasporto aggiuntivi privati, e a potenziare i controlli da parte del personale sulle banchine e nelle aree di sosta dei mezzi, garantendo l'intervento a seguito di segnalazioni puntuali e non generiche di criticità. Nessuna Regione ha chiesto nelle sedi opportune e formali di procedere ad una revisione delle linee guida, nel senso di consentire una percentuale di riempimento più bassa di quella attuale. Come Governo, siamo disponibili sempre a ricevere i contributi per il miglioramento delle linee guida, sia in ragione dell'andamento della diffusione del virus sia sulla base delle indicazioni provenienti dalla comunità scientifica. Rappresento, comunque, che i dati di utilizzo dei bus che ci hanno fornito le Regioni, che sono stati registrati a partire dallo scorso mese di settembre, si attestano attorno a meno 50 per cento (con una riduzione, quindi, del 50 per cento) rispetto allo stesso periodo del 2019, che generalmente viene rispettata anche durante le ore di punta mattutine e pomeridiane; e che la percentuale massima di riempimento dell'80 per cento consentirebbe, quindi, di soddisfare l'intera domanda di trasporto pubblico locale per lavoro e per scuola. Inoltre, in questi giorni stiamo monitorando tutti i sistemi tecnologici, testati e sperimentati dalle Regioni, per valutare di implementare ulteriormente, con l'utilizzo della tecnologia, proprio i sistemi di controllo e di monitoraggio del riempimento. Ritengo che, grazie alla fattiva collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, le Regioni, le aziende di trasporto e gli utenti, e attraverso la stretta osservanza delle attuali linee guida, che indicano anche specifiche attività e regole di comportamento, a carico sia dell'utenza che delle aziende di trasporto, la mobilità dei cittadini debba rimanere garantita come diritto per poter raggiungere i luoghi di lavoro e di studio.

mi auguro che queste vadano giustamente indirizzate e destinate, anche aumentando i controlli. È inutile, infatti, negare che i contagi sono aumentati magari proprio per una non adeguatezza dei controlli per quanto riguarda soprattutto i trasporti. Ritenendo che tutti gli operatori del settore dei trasporti abbiano bisogno di dovute misure economiche, reputo necessario non soffermarmi solo sulle linee guida. È doveroso, il Governo appronti, come ho detto prima, un piano concreto, relativo a tutto il servizio di trasporto nazionale e non solo a quello locale. La ringrazio e, come Italia Viva-PSI, restiamo disponibili a collaborare.

abbiamo già sentito anche alcune risposte del Ministro, ma io ribadisco qui alcune questioni. È evidente a tutti che ci saranno le linee guida, ma il problema c'è. Ha dimostrato esserci in modo assolutamente palese ed è stata una delle maggiori criticità emerse in questa seconda fase della pandemia.

trasporto scolastico e di 400 milioni proprio per incrementare le risorse del fondo per il trasporto pubblico locale, 300 dei quali potevano essere utilizzati per i servizi aggiuntivi di trasporto

perché come semplici utenti - soprattutto nelle grandi città - abbiamo continuato a vedere problemi, sofferenze e resse, e nessuno può venirci a spiegare

alle situazioni che si sono venute a creare. Questo è il preludio anche a un rafforzamento generale, con un piano serio -

potendolo fare in punta di diritto, per motivi politici, non è mia intenzione - e non lo sarà mai - scaricare la responsabilità su qualcun altro, nonostante le previsioni di legge. Il processo faticosissimo che questo Governo sta portando avanti per affrontare la pandemia o si affronta insieme o semplicemente non si affronta. Questo è stato lo spirito che ha improntato la nostra attività istituzionale nei confronti delle Regioni, che per la maggior parte hanno maggioranze diverse da quella di questo Governo, ma con le quali la collaborazione è sempre stata improntata alla massima professionalità, mettendo reciprocamente a disposizione tutte le competenze del Ministero e delle Regioni stesse. Credo che, in un momento così difficile, questo sia l'unico modo di lavorare di fronte alle grandi difficoltà e alle grandi criticità rispetto alle quali i cittadini ci chiedono di intervenire. La seconda puntualizzazione: ho appena provveduto a inviare alle Commissioni trasporti di Senato e Camera, cara senatrice De Petris, ricerche scientifiche (francesi, tedesche, americane) sulla verifica di come il virus si può o non si può trasmettere all'interno dei mezzi di trasporto. Tali analisi riguardano tutti i mezzi di trasporto (aerei, pullman, treni), e lì ci sono indicazioni molto interessanti perché sono analisi fatte su

Credo che i risultati di quelle analisi - che avrete la possibilità di vedere fra qualche minuto - siano particolarmente interessanti, le approfondirò nel corso del dibattito con le Commissioni riunite che si terrà alle 16,30. Inoltre, in merito alle risorse, senatrice De Petris, il decreto-legge agosto, come lei diceva, ha previsto l'immediato impiego - sui 300 milioni stanziati - di 150 milioni, di cui ad oggi sono stati utilizzati 120 milioni. Gli altri milioni sono attualmente all'esame della Conferenza unificata per la formalizzazione dell'intesa sui meccanismi di distribuzione che, a consuntivo, potranno permettere alle Regioni, quindi, di utilizzare il *plafond* messo a disposizione dal Governo di 300 milioni. In particolare, quello schema di decreto prevede che l'unico criterio definitivo di ripartizione delle risorse destinate ai servizi aggiuntivi, quindi al noleggio di pullman che possono essere messi in linea, sia quello già previsto per legge, ossia che i servizi implementati abbiano un riempimento superiore all'80 per cento. Inoltre, è stato previsto che le Regioni comunichino al MIT entro il 15 novembre i dati inerenti ai servizi aggiuntivi già resi e quelli che saranno programmati da qui a fine anno, anche per consentirci di programmare le risorse per per il 2021. Pertanto, solo dopo la data del 15 novembre potrò far conoscere al Parlamento per ogni singola Regione l'utilizzo di queste risorse. Come Governo abbiamo messo a disposizione vari strumenti, che consentono già in questa fase emergenziale di implementare, in linea con gli indirizzi della Commissione europea, le offerte di TPL e di ridurre l'impiego delle autovetture private. autovetture private. Oltre alle risorse di cui abbiamo già parlato, che sostanzialmente intervengono su circa 4.000 tratte, abbiamo anche introdotto procedure semplificate per l'affidamento delle gare - è l'articolo 1 del decreto-legge semplificazione, che lei conosce direi a memoria - e incentivato l'utilizzo dei mezzi di trasporto non di linea, ossia i taxi e gli NCC, con una norma che finanzia il *voucher* nel decreto-legge rilancio. Inoltre, da quando ci siamo insediati, abbiamo distribuito 3 miliardi, tra Regioni e città, per consentire due grandi operazioni che rifinanzieremo per i prossimi anni, ovvero il potenziamento dei progetti di trasporto rapido di massa, sui quali le città avevano già progetti maturi in termini di avanzamento, e

delle risorse messe a disposizione dal Governo e dal Parlamento. Però vorrei dirle una cosa molto chiara, signor Ministro. Verificherò queste ricerche ricerche scientifiche, ma avevamo già un livello di sofferenza non indifferente, e lei lo sa perfettamente: in tempo di pace eravamo già in grande sofferenza nelle grandi città. Io sono di Roma possiamo organizzarci un viaggio insieme, se vuole, così possiamo vedere un po' di autobus e le condizioni in cui sono. Magari uno non si prende il coronavirus, ma si può prendere qualche altra cosa. il problema dell'affollamento delle metropolitane che lei conosce perfettamente, tant'è che con lei avevamo discusso anche della metro C. Quindi, abbiamo un livello di sofferenza nelle città che in tempo di pace era già notevole. Oggi pensare che

per un piano di intervento straordinario, sapendo che prima o poi in pace ci torneremo, quindi a maggior ragione dobbiamo lavorare per un piano triennale di rafforzamento del sistema del trasporto pubblico locale.

di usare parole di verità; in parte, ne ha già fatto riferimento. Per noi del Partito Democratico, il trasporto pubblico è un tema delicato ed ha una rilevante valenza sociale. È la ragione per la quale abbiamo condiviso la scelta di non fermare il trasporto pubblico locale anche nel periodo del *lockdown*: è costato parecchio ed è una scelta che abbiamo condiviso e supportato, perché convinti dei benefici che dà alla comunità un diritto che l'Italia deve sempre garantire. In ogni caso, abbiamo condiviso anche il fatto che, sebbene il trasporto pubblico locale e il trasporto scolastico non siano di competenza dello Stato - non lo dico per polemica, perché questa è la verità lo Stato si è fatto carico di finanziare non solo le perdite dei ricavi e il rimborso dei biglietti e degli abbonamenti, ma anche i servizi aggiuntivi,

ma noi siamo qui per risolverli e non per fare polemica. Cosa è successo? Come mai questi servizi aggiuntivi sono partiti in ritardo? Inoltre pensiamo che debbano essere ancora investite risorse sul trasporto pubblico locale, che soffrirà anche

per continuare a garantire questo servizio e fare in modo che ogni polemica cessi, perché in questo momento non ne abbiamo bisogno.

come effettivamente va riconosciuto, partiamo dal presupposto di un sistema di trasporto pubblico locale profondamente differenziato, con livelli di efficienza diversi, che spesso sono diversi all'interno delle stesse Regioni, tra trasporti extraurbani e urbani, tra modalità di trasporto su ferrovia e modalità di trasporto su gomma, tra città dotate di sistemi di metropolitane e di sistemi tranviari particolarmente efficienti sul fronte ambientale, ma ancora non completamente dotati di mezzi, perché in fase di implementazione. Quindi, la pandemia accade in un momento nel quale il Governo stava sostenendo Regioni e Comuni, come ho descritto nella risposta precedente alla senatrice De Petris, proprio per potenziare tutto il sistema e per cercare di garantire un'omogeneità, sia tra Regioni che a livello intraregionale. Pensate, per esempio, alla grande attività svolta per la sostituzione e l'ampliamento del numero dei nuovi treni regionali, che è in uno stato di avanzamento molto differenziato tra Regione e Regione e questo è figlio di questioni legate alla storia di ogni singolo territorio. L'altro punto fondamentale da ricordare è che, rispetto a questa seconda riapertura totale delle attività più importanti del nostro Paese, con l'aggiunta quindi della scuola,

avremmo avuto sui mezzi un carico attorno ai 21 o 22 milioni, perché c'è già stata una riduzione naturale, legata ai temi del Covid e ad un po' di *smart working*, rimasto in campo anche durante il periodo estivo. Ad oggi le Regioni e le aziende di proprietà delle Regioni ci dicono che, complessivamente, siamo arrivati al 50 per cento in quest'ultima settimana. Da lunedì abbiamo un indicazione attorno al 50 per cento e quindi circa 15 milioni di persone. Certamente, in termini di programmazione dell'utilizzo dei fondi, abbiamo stanziato risorse sempre in accordo con le Regioni: tutto quello che sto riferendo in quest'Aula oggi e che ho riferito alle Commissioni congiunte stamane, è frutto di un accordo, peraltro verbalizzato nella Conferenza unificata del 31 agosto. 31 agosto. Ma è del tutto evidente che in alcune aree del Paese è stato più complicato fare una mappatura dei fabbisogni, perché c'è un'esigenza, negli orari di punta, radicalmente diversa dal resto della giornata. Per questa ragione, oltre a tutte le risorse che abbiamo stanziato, abbiamo chiesto fortemente a livello sia nazionale, che di istituzioni locali di attivare tavoli di *moral suasion* il più potenti possibile per continuare a garantire quanto c'è stato nei mesi di maggio, giugno e luglio di quest'anno, e cioè lo scaglionamento dei tempi di ingresso e di uscita, prima di tutto dal lavoro, e - poi - anche dalla scuola,

di trasporto o lavoro con contagio zero. Non avrei mai la presunzione di dirlo, e se leggessi uno studio di questo tipo, non ci crederei perché penso di avere un discreto realismo per non credere. se ci sono dei meccanismi di protezione e organizzazione della presenza delle persone sui mezzi di trasporto, avendo il trasporto pubblico locale il grande vantaggio di una permanenza breve degli utenti,

di consentire alle persone di esercitare il diritto alla mobilità, anche se con poche risorse (non tutti si possono comprare l'automobile). Abbiamo deciso di garantire il diritto alla mobilità proteggendo queste persone e partendo dai presupposti scientifici

del servizio, la continuità, il rimborso degli abbonamenti e la capacità di affrontare la riduzione dei ricavi. Abbiamo capito che i fondi per i servizi aggiuntivi erano pronti già dall'8 settembre scorso. Eppure, i cittadini sapranno valutare, nell'ambito delle realtà dove vivono, quando sono partiti

a lavorare perché il trasporto pubblico locale è per noi questione culturale, ma è bene che la verità sia sempre la strada maestra da seguire e la scelta migliore perché l'Italia lo merita, ancor di più in un momento di difficoltà come quello

Signor Ministro, lei sa che io sono sempre estremamente collaborativo e che Forza Italia si pone sempre come metodo in modo collaborativo e, seppure su posizioni diverse dal Governo, sempre nell'interesse generale del Paese.

uno spiegone di tre pagine dicendo di non essere d'accordo con il Governo sulle misure che sarebbero state da lì a poco prese, il Governo non gli dà importanza, va avanti, si prende le sue responsabilità e prosegue dritto.

- 120 milioni, che sono stati i primi spesi, come ci ha detto stamattina in Commissione, sono andati a finire tutti alle aziende pubbliche. pubbliche. Forza Italia ritiene che il Governo e, probabilmente, il Ministero che lei presiede siate particolarmente ostaggio del sistema della pubblica amministrazione. Lo capiamo, siete da quella parte, la difendete, ma ci sono le imprese che hanno i bus nei parcheggi e ancora non hanno visto un euro di ristoro per i *leasing* da pagare. Le segnalo che Flixbus, che fattura più di 500 milioni, in Italia non paga le tasse e il decreto che è stato precedentemente approvato società l'opportunità e la possibilità di prendere quattrini; quindi prende quattrini e noi ovviamente lasciamo le nostre aziende a secco. Per quanto riguarda il problema dei bus turistici, lo abbiamo affrontato male e nei termini sbagliati. È stato detto poco fa che Le do una notizia: una tabella del suo Ministero, che ho in mio possesso, fresca di stamani, dice che sono stati messi in servizio poco più di 1.000 autobus. Non le posso dire chi me l'ha mandata, ma mi creda, e lei sa che non le dico baggianate. È stato detto che gli autobus turistici sono grandi e non possono transitare

Oggi il Presidente del Consiglio ci chiede come mai non ci sia fiducia nel rapporto con gli italiani. Come si fa? Abbiamo avuto sei mesi per cercare di mettere a punto una serie di misure e scopriamo che il 14 settembre inizia la scuola e il 25 dicembre Natale. Mi creda: le famiglie sono ben disposte, ma ad un certo punto, quando vedono dall'altra parte un'insipienza e - non so come mai - probabilmente un'incapacità, non credo cattiva volontà, ovviamente il problema non si riesce a risolvere. Concludo facendo una battuta

più avere nuovi autobus in servizio e, di conseguenza, ancora una volta i bus turistici se ne staranno nel parcheggio. Dal decreto ristoro mancano i codici Ateco per moltissime imprese, tra cui queste, e quindi, anche questa volta, i quattrini non arriveranno. Oggi ho ascoltato parole più dure di quelle che ho pronunciato adesso io dalla sua maggioranza.

Nelle mie risposte e nella mia relazione di questa mattina in audizione presso le Commissioni riunite, alla quale lei ha partecipato, non c'è mai stato, non ci sarà, non ci vuole essere, né ho bisogno che ci sia alcuno scarico di responsabilità su altri. Quando prendiamo decisioni insieme, chi riveste un ruolo e porta questo onore e quest'onere temporaneo si assume anche la responsabilità degli altri, senza se e senza ma. Siccome tutto quello che è stato fatto fino ad ora (le cose positive e quelle negative) è stato condiviso con le Regioni, a prescindere dal colore politico, e nelle sedi istituzionali, continuerò ad andare avanti così, perché è l'unico modo modo in cui sono capace di fare il Ministro; non c'è un altro modo. Prima vengono le istituzioni, poi vengono le persone che temporaneamente ricoprono un ruolo istituzionale. Ho letto anch'io qualche distinguo, peraltro avvenuto negli ultimi minuti, da parte di alcuni assessori regionali. Me ne dispiaccio, perché casualmente, nell'ultima riunione della scorsa settimana, le medesime persone hanno detto cose esattamente opposte. Ma non conta niente,

solo una piccola soluzione in più per alleggerire la sensazione di preoccupazione che si è generata in chi utilizza il trasporto pubblico locale, sarà stata utile. E io credo che sarà così. Seconda questione: i 120 milioni di euro alle aziende di trasporto di proprietà delle Regioni sono stati utilizzati per fare le gare dei privati; quindi, queste risorse andranno ai privati,

Il fatto che l'accordo con le Regioni sia stato concluso solo alla fine di agosto non è determinato né dalla scarsa volontà politica delle Regioni, né dall'assenza di volontà politica da parte del Governo: è determinato dalla necessità di una serie di approfondimenti di natura scientifica, perché volevamo completare le linee guida sanitarie e avere il massimo della certezza

Signor Ministro, lei lo sa che non metto mai in dubbio la sua buona fede, ma le debbo chiedere di opporsi un po' di più. Capisco e conosco le problematiche interne al Governo e alla maggioranza: si opponga un po' di più. Troverà aiuto e supporto da tutto l'arco parlamentare, compresi noi, nell'interesse generale della comunità. Si confronti più spesso - come ho avuto modo di dire anche ai suoi colleghi - con il Parlamento e non faccia come il Presidente del Consiglio, che ritiene questo luogo quasi un orpello obbligatorio, in qualche modo fastidioso, costretto a parlare con noi. Le Regioni sono importanti, ma loro fanno un mestiere, mentre il Parlamento ne fa un altro. Il Parlamento è il dante causa del Governo. Siamo persone che vivono tutti i giorni il territorio, molti di noi sono imprenditori - io particolarmente nel turismo - e forse potremmo proporre

sull'approfondimento scientifico, non ci nascondiamo dietro le indicazioni del comitato tecnico-scientifico, che fa il suo mestiere e molte volte dà indicazioni che il Governo alla fine segue alla rovescia.

che è evidente a tutti che, prima o poi - neanche aspettando troppo - affonderà. Il problema è che sta affondando il Paese e non ce lo possiamo assolutamente permettere.

fra i settori maggiormente colpiti dalla crisi economica, conseguente alla crisi sanitaria Covid, vi è quello dei trasporti di massa. In particolare, le imprese del trasporto pubblico locale hanno patito perdite superiori a 1,2 miliardi di euro. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, il Governo ha stabilito un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all'80 per cento dei posti consentiti; limite da ultimo confermato anche dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, quando eravamo già in piena emergenza, perché con quest'ultimo decreto sono state chiuse molte attività. Con il decreto-legge rilancio è stato istituito un fondo a compensazione dei minori ricavi derivanti sia dal mancato utilizzo dei mezzi pubblici da parte dell'utenza, sia dagli oneri derivanti dall'obbligo di emettere *voucher* o prolungare gli abbonamenti agli utenti del servizio pubblico nel periodo non usufruito del *lockdown*. La dotazione di questo fondo, che era pari inizialmente a 500 milioni di euro, è stata aumentata di altri 400 milioni di euro con un'apposita norma contenuta nel decreto agosto. Una quota del predetto fondo di ristoro, pari a 300 milioni, può essere utilizzata per il finanziamento di servizi aggiuntivi erogati a soggetti diversi dagli affidatari dei servizi, da destinare ai servizi che nel periodo ante-Covid abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità dei mezzi. Stando ai dati in nostro possesso, dei 300 milioni stanziati per servizi aggiuntivi, al momento soltanto 120 sono stati utilizzati per finanziare - dato oggi da lei confermato - 4.000 corse aggiuntive al giorno, concentrate nelle direttrici ad alta densità e nelle grandi aree metropolitane; ciò perché la norma prevede l'adozione di un decreto di riparto di tali risorse che al momento non risulta ancora emanato.

Tutte le misure, comunque, sono risultate inefficaci per la riduzione del sovraffollamento dei mezzi e per la diffusione del contagio. È vero anche che non esistono studi che ci dicano che la diffusione dei contagi avviene all'interno dei mezzi pubblici, ma penso sia sotto gli occhi di tutti perché, nel momento stesso in cui chiudiamo i bar, i ristoranti e altre attività come le palestre, non vedo perché all'interno dei mezzi pubblici non ci si possa comunque contagiare. *(Applausi)*. Chiediamo quindi al Ministro quali azioni da oggi intenda intraprendere e attivare con la massima urgenza. Non possiamo aspettare - come diceva prima - il 15 novembre. Siamo in emergenza.

dell'imminente riapertura delle scuole che si sarebbe poi realizzata il 14 settembre, nella quale veniva chiesto che venisse garantito il riempimento dei mezzi pubblici al

abbiamo trovato, insieme al comitato tecnico-scientifico, la possibilità di dare una risposta ai fabbisogni senza arrivare al riempimento totale dei mezzi, con l'autorizzazione al riempimento all'80 per cento e con tutta una serie di misure sanitarie che caratterizzano specificamente solo il trasporto pubblico locale. Inoltre, nel 2020 abbiamo stanziato 900 milioni in più, oltre a quelli di cui già le Regioni sono titolari per il trasporto pubblico locale, per garantire la minore bigliettazione, e cioè la copertura della stragrande maggioranza dei minori ricavi. Siamo arrivati a un accordo all'unanimità non solo sulle linee guida, ma anche sull'utilizzo e i criteri dei 300 milioni. E qui mi soffermo, onorevole senatrice; onorevole senatrice; 150 milioni di questi 300 sono automaticamente assegnati e non hanno bisogno di alcun atto amministrativo di assegnazione. Ne sono già stati utilizzati 120 per implementare, con tutto quello che le aziende hanno ritenuto essere necessario, le corse su gomma. Non sfuggirà a nessuno dei presenti che le corse su treno o comunque sulle metropolitane non sono così facilmente implementabili; si può arrivare a un massimo della capienza della frequenza, ma non si può andare in un autosalone ad acquistare un treno. Tant'è vero che abbiamo molte Regioni che hanno in ordine il rinnovo dei mezzi, ma con termini di dodici, tredici e diciotto mesi. Detto questo, gli altri 150 milioni - a cui forse faceva riferimento con la sua citazione legata alla distribuzione alle Regioni - con il con il decreto del Ministro sono già all'attenzione della Conferenza, di cui stiamo attendendo il parere. La proposta che abbiamo fatto alla Conferenza è quella di distribuirli con gli stessi criteri con cui sono stati assegnati i precedenti 150

dei percorsi, urbani o extraurbani, è bene concentrarsi sui percorsi già stressati, perché hanno un numero importante di passeggeri e di persone. Un'ultima cosa mi sono dimenticata di dire nelle mie risposte: dopo vari mesi di sperimentazione che abbiamo chiesto ad alcune società del trasporto pubblico in varie parti d'Italia, sono arrivate a definizione alcune applicazioni tecnologiche che potranno essere utili per migliorare la qualità del servizio. Per questo domani si terrà la riunione di un tavolo tecnico che ho istituito, alla presenza del ministro Pisano e degli uffici del Ministro per l'innovazione per fare una valutazione tecnica su quali sono le sperimentazioni andate meglio ed eventualmente metterle a disposizione di tutte le Regioni e le aziende di trasporto pubblico locale.

Operazione verità: solo l'8 settembre, con il decreto-legge n. 111 dell'8 settembre 2020, avete messo in campo 300 milioni per i servizi aggiuntivi. Una settimana prima dell'inizio delle scuole: alla faccia della programmazione!

Così come è giusto riconoscere il fatto che 300 milioni, su 105 miliardi utilizzati in scostamento per affrontare l'emergenza, sono un po' pochi per 20 Regioni; me lo faccia dire onestamente.

Quindi le Regioni non potevano usarli per fare chissà quali tipi di servizi; lei sa che i bus turistici si possono utilizzare non nelle linee urbane, ma solo nelle linee extraurbane.

urbane, quelle a maggior densità - stiamo parlando di città come Milano, Torino, Roma e così via - perché il ministro Gualtieri non ha ad oggi ancora messo la firma. *(Applausi)*. Sono passati quattro mesi. mesi. Per chiudere, signor Ministro, più che continuare a scaricare sulle Regioni, dicendo che avete fatto il possibile per aumentare le corse, date l'impressione di essere un Governo a fine corsa.

con la presente interrogazione chiediamo spiegazioni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sui contenuti del piano economico-finanziario (PEF) con cui si definiscono interventi, investimenti e tariffe all'interno del rapporto con il concessionario Autostrade per l'Italia SpA Il 22 settembre 2020 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) la proposta di aggiornamento del suddetto Piano economico-finanziario, su cui lo scorso 14 ottobre l'Autorità ha espresso un parere estremamente critico, rilevando che «il Piano economico-finanziario (...) presenta alcune significative difformità applicative (...) potenzialmente idonee a riflettersi anche sui livelli tariffari applicabili all'utenza» che il Piano, ora come ora, prevede una variazione tariffaria media annua dell'1,75 per cento, che invece, secondo le stime dell'ART, dovrebbe valere lo 0,87 Altra censura dell'Autorità è legata ai costi delle manutenzioni incrementali, cioè quelle aggiuntive da dover fare per compensare le mancanze di gestione degli anni precedenti. Secondo il parere, l'inclusione di tali interventi in tariffa va attentamente valutata dal Ministero delle infrastrutture Infine, l'Autorità contesta anche l'inclusione in tariffa di un onere correlato agli effetti economici innescati dall'emergenza Covid-19, mentre il sistema tariffario dell'ART prevede il trasferimento del rischio tariffario soltanto in capo al concessionario. Alla luce delle evidenze dell'Autorità, appare più concreta la volontà di Autostrade per l'Italia SpA di incrementare notevolmente i propri profitti, a scapito degli utenti destinatari dei pedaggi maggiorati. Tale scenario è assolutamente contro corrente rispetto all'azione governativa in essere. È appena il caso di ricordare che, a seguito della tragedia del ponte Morandi, il Governo ha dapprima avviato una procedura amministrativa per valutare la revoca della concessione; successivamente questa iniziativa è sfociata nella delicata trattativa, attualmente in corso con Cassa depositi e prestiti, a ricondurre il concessionario a una gestione pienamente coerente con gli interessi pubblici coinvolti, attraverso la partecipazione della medesima Cassa depositi e prestiti, controllata dal Ministero dell'economia e dei trasporti sa, questa complessa e delicata trattativa punta a rilevare da Atlantia SpA, *holding* controllata dalla famiglia Benetton, la partecipazione in Autostrade per l'Italia, per permettere l'ingresso di una cordata di investitori guidati da Cassa depositi e prestiti. La stessa trattativa rischia tuttavia di essere irreversibilmente alterata da un Piano economico-finanziario che, garantendo eccessivi vantaggi all'attuale concessionario, è potenzialmente in grado di influire negativamente sul prezzo di cessione.

soprattutto in questa fase di delicate trattative con Cassa depositi e prestiti, e per evitare che si creino irreversibili effetti sui termini, anche e soprattutto economici, della suddetta trattativa.

dall'agosto del 2018 nei confronti di Autostrade per l'Italia SpA a seguito del tragico evento del crollo del ponte Morandi, è stata poi sospesa nel mese di luglio 2019, a seguito della richiesta, che la società stessa ha fatto al Ministero, di avviare una fase finalizzata a un accordo transattivo e a una modifica radicale della convenzione, maggiormente rispondente all'interesse pubblico e depurata da pattuizioni sbilanciate a favore del concessionario. La fase per la verifica di un possibile accordo transattivo, che è stata avviata proprio dal precedente Governo, è stata da me poi proseguita a settembre 2019, a seguito di una specifica decisione dell'Esecutivo. In particolare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha portato avanti un confronto molto duro poi alla valutazione del Governo; tutto ciò nel rispetto del principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa, anche a seguito delle risultanze della commissione che aveva fatto una verifica sulle conseguenze dell'attuazione della revoca, al fine esclusivo di

transattive trasmesse e giunte all'esito di una lunga e complessa valutazione di tutte le problematiche tecnico-giuridiche e di un minuzioso confronto tra gli uffici del mio Ministero, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, avviando l'*iter* previsto dalla legge per la formale predisposizione di una transazione. È dunque nell'ottica di tale soluzione concordata, volta a garantire la piena realizzazione dell'interesse pubblico connesso all'esigenza di consentire all'utenza di continuare a fruire dell'infrastruttura, di salvaguardare i livelli occupazionali, di effettuare nuovi e consistenti investimenti e di tutela dei risparmiatori, che deve essere oggi considerato il piano economico-finanziario (PEF) che è stato presentato da Aspi, non Nell'evidenziare che il MIT e le altre amministrazioni coinvolte hanno costantemente rappresentato alla società la necessità di sviluppare la proposta del PEF recependo puntualmente tutte le indicazioni della nuova regolazione tariffaria introdotta dall'Autorità di regolazione dei trasporti, ricordo che l'approvazione del PEF da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia, segue precise regole procedurali, tra cui l'acquisizione del parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Le osservazioni formulate dall'Autorità sulla proposta di PEF di Aspi sono attualmente oggetto di specifici approfondimenti, che saranno ovviamente resi noti non appena definiti, ma hanno contenuti per molti versi difformi da quanto ho appena sentito. Concludo comunque tranquillizzando gli onorevoli interroganti ed evidenziando che questo snodo procedurale risponde unicamente alle regole tecniche di carattere economico-finanziario, oltre che trasportistico ovviamente, ma non influenza la trattativa riguardante gli impegni di Aspi e di Atlantia sul futuro assetto societario, che tra l'altro non è gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in relazione alla quale comunque vi posso riferire che Cassa depositi e prestiti ha confermato al Governo che tutte le interlocuzioni si svolgono sulla base di criteri competitivi e di prassi correnti di mercato e, quindi, non riconducibili alla vicenda del PEF. finestra") *(M5S)*. Signor Ministro, siamo evidentemente preoccupati perché siamo di fronte a una questione a dir poco delicatissima. Sarebbe importante, signor Ministro, se riuscissimo ad interloquire.

evidentemente e oggettivamente preoccupati, perché siamo di fronte a una questione delicatissima, intrecciata: da una parte abbiamo le nuove tariffe e i nuovi termini della concessione, il piano economico-finanziario che il MIT, quindi lo Stato concedente, fa con Aspi; dall'altra, abbiamo abbiamo una delicatissima trattativa che un soggetto pubblico, in questo caso Cassa depositi e prestiti, sta portando avanti per far entrare lo Stato e far sì che si sostituisca a quell'interesse privato e a quella parte societaria maggioritaria del concessionario che si è comportata oggettivamente malissimo nella gestione dei 6.000 chilometri

perché conta svariati miliardi in più di entrate per il concessionario privato, rispetto a quanto dovrebbe prevedere la regolamentazione, nata in conseguenza di un articolo del cosiddetto decreto Genova, che ha portato l'Autorità di regolazione dei trasporti a creare il nuovo modello tariffario. Il nuovo modello tariffario significa semplicemente una cosa: pedaggi più bassi, manutenzione più alta, più sicurezza e meno extraprofitti per il concessionario.

decreto Genova, modello tariffario ART, e in quella legge le manutenzioni devono aumentare; chi non le fa paga la penale, che abbiamo previsto noi dopo la tragedia del ponte Morandi. Deve aumentare la sicurezza e i pedaggi devono diminuire. Va detto loro semplicemente questo.

un abuso della cosa pubblica, che in questo caso era l'autostrada. Forza Ministro, quindi, faccia vincere i cittadini italiani e l'interesse pubblico sulla bramosia di profitto di questi colossi, che ha vinto invece contro lo Stato e contro i cittadini per decine di anni. Significa che, che, quando andremo al casello a pagare il pedaggio, pagheremo un po' di più e vedremo qualche cantiere in più, che renderà più sicure le nostre autostrade.

per metterle al corrente dell'intenzione di ricorrere al Fondo di integrazione salariale (FIS) dal 2 al 15 novembre per i dipendenti a tempo determinato e indeterminato di tutte le unità produttive della fondazione, fino al 100 per cento dell'orario di lavoro. Ciò si traduce in una decurtazione dello stipendio pari al 40 per cento per le maestranze contrattualizzate. Orbene, nei circa quattro mesi di *lockdown* le 14 fondazioni lirico-sinfoniche italiane, nove delle quali - com'è noto - sono monitorate da un commissario straordinario di Governo, hanno sospeso attività e spettacoli. Ne sono derivati sia un mancato incasso al botteghino per gli spettacoli annullati, sia un risparmio sui costi di produzione legati ai compensi degli artisti, degli ospiti e agli allestimenti scenici, oltre che agli stipendi tagliati di cui dicevo. Poiché le fondazioni hanno incassato per l'anno in corso contributi dallo Stato e dagli enti locali, il risparmio dovuto alla sospensione degli spettacoli, peraltro incrementato dalla mancata contrattualizzazione dei tanti lavoratori precari stagionali e intermittenti, che da tempo riempiono gli organici delle fondazioni, in attesa della piena applicazione del decreto-legge n. 59 del 2019, è ampiamente superiore ai mancati incassi di botteghino. Il margine di produzione sarà quindi positivo per tutte. In queste condizioni, l'eventuale ricorso al FIS per i dipendenti da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche, per quanto non illegittimo, appare quantomeno inopportuno. Qual è la *ratio* di questa scelta? Impiegare quelle risorse per la cassa integrazione senza reali necessità economiche e produttive, poiché il Ministero per ha ribadito - da ultimo proprio il 27 ottobre - la possibilità di allestire spettacoli da mandare in scena ad esempio in *streaming*, significa penalizzare le maestranze contrattualizzate e sottrarre quelle risorse alla priorità del momento, che è la tutela dei lavoratori dello spettacolo meno protetti, intermittenti, stagionali, precari da sempre, che non lavorano da marzo a causa della pandemia. Le fondazioni, avendo ricevuto integralmente i finanziamenti preventivati - lo ripeto - dovrebbero quindi ricorrere alla certificazione economico-finanziaria redatta dal collegio dei revisori dei conti, che attesti la necessità di detti sussidi allo scopo di evitare una perdita di esercizio. Mancando tale documentazione, ritengo difficile che possano evitare uno scandalo all'atto della presentazione dei bilanci consuntivi per avere chiesto sussidi statali in presenza di ingenti utili e lo scandalo ovviamente coinvolgerebbe anche chi quei sussidi ha concesso. La priorità - torno a dirlo - sono

è la richiesta di finanziamenti per gli investimenti sulla rete ferroviaria italiana in Sardegna. Come già noto, uno dei problemi principali della logistica sarda è la sua situazione ferroviaria. Difatti, la rete ferroviaria sarda è caratterizzata da bassa velocità e scartamento ridotto. In tutta Italia, da Nord a Sud, si progettano e si realizzano le reti ferroviarie di alta velocità e capacità per passeggeri e merci, il doppio binario, l'elettrificazione diffusa: ovunque, tranne che da noi. Dobbiamo forse sentirci in colpa perché viviamo su un'isola? Secondo l'istituto Tagliacarne, che misura il divario infrastrutturale, la nostra è la peggiore rete ferroviaria italiana. Una nota positiva c'è. Proprio qualche giorno fa, è stato inaugurato il nuovo treno Swing, destinato a poche tratte. Subito sono nate le preoccupazioni, perché non è certo che i treni di questo tipo abbiano la possibilità di percorrere tratte ferroviarie obsolete, con conseguenze di servizi inaccettabili e rischiosi. Con questa situazione, credo sia indispensabile garantire alla Sardegna i finanziamenti necessari per il superamento dell'attuale svantaggio competitivo, al pari di quanto stanziato per molte altre Regioni italiane da Nord a Sud. Nel maggio 2020 è stato sottoscritto un accordo quadro tra la Regione Sardegna e RFI, in attuazione del disegno di legge n. 112 del 2015, strumento di coordinamento e pianificazione, oltre che programmatorio, che migliorerebbe la qualità del servizio ferroviario. La Regione Sardegna, in accordo con il gruppo FS, è impegnata a potenziare e rendere efficiente il trasporto pubblico. Ha previsto investimenti per rinnovare e velocizzare le linee ferroviarie del gruppo su tutta l'isola. Il punto è il seguente: gli interventi per lo sviluppo infrastrutturale e tecnologico, pur condivisi nell'accordo, non trovano copertura finanziaria, se non in minima parte. Intercalo un dato interessante. Secondo il rapporto Pendolaria di Legambiente, negli ultimi anni la Sardegna ha incrementato il numero di passeggeri del 18 per cento. Questo ci fa capire ancora di più quanto siano necessari un miglioramento e un incremento dell'efficienza dei trasporti ferroviari. Tra gli investimenti da finanziare, vanno ricompresi l'elettrificazione della rete ferroviaria a sud di Oristano, incluso tutto il Sulcis; il raddoppio del binario tra le località di Villamassargia e Decimomannu, nonché tra San Gavino e Oristano; il potenziamento il potenziamento della linea ferroviaria Macomer-Olbia, di rilevanza strategica per il futuro della nostra isola; ma soprattutto il collegamento con il porto e l'aeroporto di Olbia. Chiedo, a nome di tutti i sardi, una cosa molto importante: il Governo intervenga con non meno di 900 milioni di euro, cifra minima se si vuole realizzare una reale opera di svecchiamento della rete, e con almeno 100 milioni di euro per interventi sulle opere di alta velocizzazione. *(Applausi)*.